Signor Presidente, onorevoli senatori, l'Italia e la Libia sono accomunate da vicinanza geografica, da legami storici e culturali, da forte complementarità tra le rispettive economie e sentimenti soprattutto di profonda amicizia tra i due popoli. Questi legami affondano le loro radici nella particolare qualità del dialogo instauratosi nel tempo tra le società e tra i popoli dei nostri due Paesi e sono stati alimentati dal gesto di riconciliazione che l'Italia ha voluto compiere, cancellando le recriminazioni lasciate dal passato coloniale. Questi sentimenti di amicizia con il popolo libico ci avevano spinti a favorire con tutte le nostre forze una soluzione pacifica alla crisi. I nostri atti, sin dal primo momento, prima ancora della risoluzione n. 1973, sono stati tesi all'unico obiettivo di impedire che quella che è stata chiamata la «primavera del Mediterraneo» fosse soffocata nel sangue. abbiamo anche sperato che il colonnello Gheddafi potesse scegliere la via dell'esilio, ipotesi evocata da più parti per evitare il massacro dei civili. Abbiamo perciò condiviso prima le sanzioni della risoluzione n. 1970 e poi le più drastiche misure previste dal capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite. Non si tratta affatto, onorevoli senatori, di fare la guerra, ma di impedire la guerra e le sue nefaste conseguenze. Si tratta di portare aiuto a chi è in balia di un'offensiva bellica indiscriminata. E, per portare questo aiuto, è necessaria la forza, il diritto e il dovere di proteggere che le Nazioni Unite hanno solennemente sancito. La risoluzione n. 1973 rappresenta perciò lo sbocco di una graduale azione diplomatica della comunità internazionale. Con la sua adozione e con il suo mancato rispetto da parte del regime libico la pagina è stata voltata. Il regime si è posto definitivamente fuori dalla cornice di legalità internazionale. La risoluzione ha confermato l'obiettivo primario della protezione della popolazione civile adottando più stringenti misure, come l'istituzione di una zona di divieto di sorvolo. La decisione, come voi sapete, è anche espressione di richieste precise della Lega araba e risponde in termini politici all'appello del Consiglio nazionale libico di transizione di Bengasi. Il Governo ha costantemente tenuto informato il Parlamento sugli sviluppi della crisi. Abbiamo condiviso con il Parlamento l'intenzione di partecipare all'intervento in attuazione della risoluzione dell'ONU n. 1973. Abbiamo ottenuto il via libera delle Commissioni affari esteri e difesa di entrambe le Camere. Ecco perché, su tali basi, abbiamo assicurato la nostra partecipazione a pieno titolo alle operazioni che sono state avviate. In tale quadro di condivisione delle responsabilità, l'Italia sta dando e darà il proprio contributo all'applicazione della risoluzione n. 1973, nel puntuale rispetto dei limiti da essa definiti. Abbiamo garantito l'utilizzo delle basi militari sul territorio italiano e l'impiego di uomini e mezzi (aerei e navali) delle nostre Forze armate; la nostra azione è condotta in stretto coordinamento con i *partner* internazionali e in contatto con i diversi attori con i diversi attori regionali. Onorevoli senatori, l'azione militare serve ad evitare danni gravissimi. Per questo ci siamo e ci saremo con piena dignità e faremo valere i principi assoluti di solidarietà e di civiltà, quando li sentissimo messi tra parentesi o addirittura calpestati. Ma restiamo anche convinti del fatto che la soluzione della crisi passi attraverso l'avvio del dialogo nazionale, di un autentico processo costituente che coinvolga le componenti politiche, sociali e tribali della Libia. Un dialogo, questo, ed una soluzione politica con una sola precondizione, che l'intera comunità internazionale, e con essa l'Italia, ha posto: l'abbandono del potere da parte del colonnello Gheddafi. A pochi giorni di distanza dall'avvio delle operazioni, il Governo torna quindi in Parlamento per informarlo degli ultimi sviluppi. Vogliamo condividere l'impegno volto Grazie per ribadire la volontà di ripristinare con la Libia del dopo Gheddafi quel rapporto preferenziale che è a nostro avviso idoneo a tutelare i nostri interessi nazionali, compresi quelli economici. È un impegno - spero, onorevoli senatori - che potrà mostrare unite le istituzioni e la politica dell'Italia, in nome dell'interesse superiore generale del Paese. Approvata quindi la risoluzione, era necessario partire con un'azione urgente che scongiurasse in via temporanea - ovviamente un'azione temporanea, ancorché urgente - un massacro di civili. Superata questa primissima fase, dobbiamo ora tornare alla fisiologia, dobbiamo tornare alle regole: un'unica catena di controllo e comando assicurata dalla NATO. Nel contempo, siamo convinti della necessità di coinvolgere attivamente l'Unione europea, specialmente per gli aspetti umanitari della crisi. Una forte consultazione politica, uno stretto coordinamento operativo faranno la differenza nella realizzazione delle operazioni prescritte dalla risoluzione, garantendo efficienza, coerenza, condivisione delle scelte politico-strategiche. Le conseguenze delle operazioni, onorevoli senatori, ricadono su tutti i *partner* e dobbiamo dunque evitare il rischio di essere corresponsabili di azioni non volute. Ecco perché dobbiamo trovare formule adeguate per coinvolgere politicamente un numero più ampio di Paesi, a cominciare dai *partner* del mondo arabo. Un comando e controllo garantito da un'organizzazione dalla consolidata esperienza, qual è la NATO, assicura coesione ed efficacia della coalizione. Questa nostra posizione, autorevolmente sostenuta anche dal presidente Napolitano, è stata condivisa da gran parte degli alleati. Su di essa, come sapete, gravava una riserva francese. Nella notte, a seguito di una conversazione telefonica tra il presidente Obama e il presidente Sarkozy, quest'ultimo ha accettato il passaggio ad una fase che riconosca il ruolo chiave della NATO per l'attuazione della risoluzione n. 1973. A questa soluzione abbiamo contribuito con un atteggiamento fermo. Io stesso avevo potuto esprimere, lunedì scorso a Bruxelles, la posizione secondo cui, qualora non fosse stato raggiunto un accordo tra i Paesi alleati sul coordinamento NATO, l'Italia avrebbe dovuto anche considerare l'ipotesi di riassumere una responsabilità nazionale per le proprie attività. Ed ecco allora che una netta preferenza per il quadro NATO si è delineata. Essa era stata espressa anche dai Paesi arabi pronti a partecipare alle operazioni, come ad esempio gli Emirati arabi uniti ed il Qatar. Ho avuto occasione proprio ieri di ascoltare in una conversazione l'opinione del Ministro degli esteri emiratino, il quale mi ha detto che l'assenza di un coordinamento NATO è stata uno dei fattori che hanno rallentato il processo di adesione degli Emirati alle operazioni. Egli ha anche smentito l'asserita contrarietà dei Paesi del Golfo all'attribuzione alla NATO del ruolo chiave che noi auspicavamo. La stessa Turchia, come sapete, ha poi accettato con equilibrio questa soluzione in quanto membro della NATO, e Kuwait e Giordania, come voi certamente saprete, hanno deciso di fornire appoggio logistico all'operazione. Sempre in ambito NATO, l'Italia ha chiesto e ottenuto che l'embargo sulle armi sia attuato anche tramite un'operazione navale di pattugliamento delle acque internazionali, e l'Italia svolgerà un ruolo cruciale con il comando dell'operazione da Napoli con un ammiraglio italiano. Quanto al ruolo attribuito all'Unione europea, il Consiglio dei ministri degli esteri, lunedì scorso, ha confermato l'obiettivo primario della protezione delle popolazioni civili e del sostegno alle loro aspirazioni democratiche. Abbiamo espresso la nostra determinazione ad agire d'intesa con i *partner* internazionali e in particolare con i membri della Lega araba. L'Unione europea continuerà a fornire assistenza umanitaria ai civili vittime delle violenze. L'Unione europea può fornire sostegno materiale, incluso l'utilizzo di assetti della protezione civile europea, per le iniziative internazionali di soccorso e di evacuazione coordinate sotto l'egida sotto l'egida delle agenzie dell'ONU e nel rispetto delle linee guida delle Nazioni Unite sull'uso dei mezzi di difesa civile e militare. Abbiamo inoltre invitato l'Alto rappresentante - ed è questa anzitutto una richiesta italiana - a sviluppare la pianificazione di un'operazione di assistenza umanitaria e di protezione civile anche attraverso l'impiego di mezzi navali: un'azione europea da condurre in stretto coordinamento con l'ONU, con la NATO, con le altre organizzazioni regionali ed i Paesi vicini coinvolti. Un'operazione, com'è ovvio, anche di forte deterrenza, questa europea, nei confronti delle organizzazioni criminali dedite al traffico di esseri umani. La pianificazione dell'azione sarà condotta in tempi rapidi; la valuteranno gli Stati membri dell'Unione europea entro la fine di questa settimana. E l'Italia ha messo a disposizione il quartier generale operativo per l'attuazione di questa missione europeo-mediterranea. Un'offerta apprezzata richiesta, ha inserito proprio lunedì, nel punto 7 della risoluzione, il principio di solidarietà e l'impegno verso i Paesi, come l'Italia, più esposti all'impatto dell'immigrazione illegale. Nel quadro delle misure adottate dall'ONU, siamo stati e rimaniamo impegnati a dare attuazione alle sanzioni finanziarie, comprese quelle decise dall'Unione europea.

2 miliardi, fino al limite massimo raggiunto negli Stati Uniti di beni congelati per 30 miliardi. Abbiamo anche sottolineato l'esigenza che i bisogni primari del popolo libico siano tenuti in considerazione con specifiche clausole di salvaguardia umanitaria. Il Consiglio europeo di domani, 24 marzo, adotterà poi le sanzioni sui prodotti petroliferi, in particolare nei riguardi della compagnia petrolifera libica (la sua compagnia di Stato) e delle sue sussidiarie.

il colonnello Gheddafi aveva minacciato di sostituire gli acquirenti europei con quelli di altri Paesi. Ora non può più farlo precludendo ad ogni potenziale acquirente, al mondo, di comprare petrolio libico, siamo ormai tutti tutelati nella medesima maniera. Non c'è più il rischio che che le compagnie europee siano scavalcate da parte di società concorrenti, perché tutti i Paesi membri delle Nazioni Unite sono tenuti a rispettare l'embargo, e ciò anche in ossequio al principio di non alterare, con misure, ovviamente, illegali, la concorrenza internazionale. Non è allora fondata la tesi secondo cui i contratti delle nostre imprese sarebbero stati meglio tutelati in caso di nostro mancato intervento. Le sanzioni internazionali contro il regime li avrebbero comunque svuotati di ogni efficacia, ed analogo ragionamento sarebbe valso nel poco realistico caso in cui Gheddafi dovesse, alla fine, prevalere. In ogni caso le sanzioni continuerebbero a dispiegare i loro effetti e renderebbero inefficaci e inapplicabili i contratti firmati. Ciò non toglie, ovviamente, che occorre continuare ad operare per tutelare, per il futuro della Libia, le posizioni contrattualmente acquisite dalle imprese italiane sul mercato libico. Faremo valere la piena efficacia dei contratti quando la loro vigenza non sarà più bloccata dal regime sanzionatorio. Lo stesso Consiglio transitorio di Bengasi ha assicurato di voler adempiere a quei contratti, dicendosi convinto del fatto che il rispetto delle libertà economiche dello Stato di diritto costituisce un aspetto cruciale delle rivendicazioni libiche, di quella che oggi è l'opposizione libica e di quella che noi speriamo sarà domani la nuova Libia. Nel frattempo, le imprese europee, impossibilitate ad onorare i contratti in ragione delle sanzioni ONU, trovano oggi, proprio in un regolamento dell'Unione europea che abbiamo recentemente adottato, una misura importante di tutela. È il regolamento n. 204 del marzo 2011, il quale preclude eventuali azioni legali per inadempimento contrattuale. Il regolamento europeo prevede modalità per assicurare i pagamenti dovuti alle imprese europee in base a contratti precedenti ed eseguiti prima dell'entrata in vigore delle sanzioni. Vi è una questione delicata che il Parlamento ha posto, quella del Trattato bilaterale. Il Trattato bilaterale è stato evocato per chiedere al Governo una valutazione sulla condizione giuridica in cui esso si trova. Da un punto di vista giuridico, onorevoli senatori, l'Italia opera nel rispetto degli obblighi di diritto internazionale. Fino all'adozione delle risoluzioni dell'ONU, l'Accordo di amicizia poteva considerarsi di fatto sospeso alla luce dei principi generali in materia di estinzione e sospensione dei trattati internazionali. Questa era stata la posizione del Governo fino all'adozione delle risoluzioni dell'ONU. Ma il quadro legale è oggi cambiato. Ora l'Italia è chiamata a rispettare la risoluzione n. l'articolo 103 della Carta dell'ONU afferma la prevalenza assoluta ed automatica degli obblighi della Carta su quelli assunti dagli Stati membri con qualsiasi altro accordo, internazionale o bilaterale. Siamo quindi tenuti ad adempiere decisioni vincolanti del Consiglio di sicurezza. Ne discende, onorevoli senatori, la sospensione, di diritto e non più di fatto, automatica degli obblighi del Trattato bilaterale, la cui applicazione sarebbe in contrasto con la risoluzione n. 1973. Tale interpretazione, del resto, è desumibile dallo stesso Accordo che riconosce la centralità delle Nazioni Unite e impegna le parti al rispetto della legalità internazionale. Dobbiamo considerare, inoltre, che i soggetti di diritto internazionale non sono i Governi ma sono gli Stati, considerazione che ci spinge a guardare al futuro delle nostre relazioni bilaterali e all'interesse a mantenere in vita il Trattato, ancorché sospeso di diritto in via automatica, per conservare in prospettiva un rapporto preferenziale con la Libia del dopo Gheddafi. Nell'ambito dell'intervento internazionale va privilegiata l'assistenza umanitaria. L'Italia è pronta all'azione intrapresa verso la Libia, verso la Tunisia, verso l'Egitto, con un forte coinvolgimento delle organizzazioni internazionali. Signor Presidente, l'Italia è stato il primo Paese che ha portato aiuti umanitari a Bengasi. *(Applausi)*. Con due navi italiane sono arrivate 90 tonnellate di materiale: cibo, *kit* medicinali e beni di prima necessità per gli ospedali. È una testimonianza concreta, al di là dei facili proclami spesso non seguiti dai fatti, di una vicinanza reale ai bisogni e alle richieste del popolo libico. Vogliamo continuare ad essere protagonisti nell'aiuto umanitario a quel popolo che soffre. Ma vi è anche un altro aspetto estremamente delicato: quello dell'immigrazione. Molti avevano tacciato come allarmistica la previsione di massicci afflussi di migranti. Ebbene, dalla Tunisia abbiamo visto un forte afflusso di migranti, che ci ha indotto a chiedere con forza che la solidarietà europea per fronteggiare l'emergenza migratoria sia riaffermata in modo chiaro. Da gennaio, 15.000 ed oltre immigrati clandestini sono arrivati in Italia. Non parlo delle condizioni di disagio di Lampedusa, ma della condizione di tutti i centri che si trovano in regioni italiane. La concreta possibilità che nuovi, ed anche superiori, flussi provengano presto dalla Libia impone in ogni caso una strategia in chiave europea. Abbiamo avanzato alcune richieste: maggiore cooperazione dell'Unione con i Paesi della sponda Sud, anche per garantire la sicurezza delle frontiere; gestione europea dei flussi sulla base di una condivisione effettiva degli oneri tra tutti gli Stati membri; definizione, infine, di un sistema unico di asilo europeo e maggiore collaborazione nella identificazione dei cittadini non comunitari. Questi principi sono stati raccolti nelle conclusioni del Consiglio europeo dell'11 marzo scorso (un Consiglio europeo straordinario chiesto anzitutto dall'Italia) e confermati dai Ministri degli affari esteri il 21 marzo scorso. In conclusione, onorevoli senatori, credo si debba dire come l'Italia ed il Governo italiano vedono la prospettiva politica per il futuro della nuova Libia. La dimensione politica e quella del partenariato rappresentano la prospettiva su cui dobbiamo impegnarci maggiormente. Uno dei punti più importanti della risoluzione è l'invito a promuovere un dialogo nazionale di riconciliazione. Spetta all'Unione europea, all'ONU, alla Lega araba e all'Unione africana facilitare quel dialogo, favorendo il coinvolgimento dei gruppi tribali di cui la Libia è composta. far funzionare ed attuare da subito il cessate il fuoco e la *no-fly zone*; ciò vuol dire fermare le violenze e creare le condizioni affinché il dialogo di riconciliazione nazionale possa davvero svilupparsi. Credo che sia l'ONU a dover verificare sul terreno il cessate il fuoco, e su questa base una fase politica si potrebbe aprire. L'Italia ha aperto da subito un canale diretto con Bengasi: abbiamo contatti costanti. Io personalmente ne ho avuti con il Presidente del Governo provvisorio libico, l'ex ministro della giustizia Jalil. Abbiamo riaperto a Bengasi il consolato italiano; siamo regolarmente informati dei rapporti con le autorità locali; esponenti del Consiglio di Bengasi sono venuti a Roma a rappresentare richieste e prospettive: l'obiettivo della riconciliazione e anche quello dell'integrità territoriale del Paese. Non vogliamo una Libia divisa in due; essa non sarebbe nell'interesse del popolo libico, e lo stesso comitato di Bengasi ha sempre mostrato forte contrarietà a questa prospettiva. Lavoreremo senza paternalismi per favorire una transizione democratica di un Paese che è al centro del Mediterraneo e di vitali interessi nazionali Concorreremo portando un contributo originale dell'Italia all'incontro che l'Unione africana ha promosso venerdì prossimo ad Addis Abeba con l'Unione europea, l'ONU e la Lega araba per riflettere sulle prospettive politiche del futuro della Libia. Vogliamo lavorare su una vera integrazione euromediterranea di tutti i Paesi della sponda Sud: una stagione politica che, nell'avvicinarsi della vera democrazia e di una stagione di diritti, preservi i popoli dalle pericolose tentazioni di influenze radicali o fondamentaliste. In conclusione, signor Presidente, siamo impegnati con piena responsabilità, leali alla coalizione e al rispetto della legalità internazionale. Oggi non portiamo la guerra in Libia; siamo e saremo ancora di più attenti alla popolazione civile, all'uso della forza strettamente conforme alle regole dell'ONU e alla ricerca di una riconciliazione nazionale che, dopo il regime, offra al popolo libico prospettive di prosperità e di autentica libertà.

che la comunicazione del ministro Frattini sia largamente esaustiva anche di molti argomenti che avrei potuto

Grazie sufficiente rilievo è quello della straordinaria accelerazione dei tempi operativi che è avvenuta in questa vicenda come mai era successo nelle pur molteplici crisi internazionali degli ultimi anni. Dal momento in cui si è posta l'eventualità di un intervento internazionale al momento in cui è poi arrivata una risoluzione, fino al momento in cui la risoluzione è diventata poi operativa, è passato un tempo così breve come mai era capitato in precedenti occasioni. Non ci interessa tanto individuare esattamente i fattori che hanno determinato questa accelerazione, quanto capire cosa questo ha comportato. Va comunque detto quali sono state le ragioni di questa accelerazione: essa da un lato ha risposto all'esigenza di fermare i combattimenti in atto in quella che era divenuta una vera e propria guerra tra le fazioni contendenti di una Libia spaccata in due, con gravissime ripercussioni sulla popolazione civile; d'altro lato ad influenzare l'accelerazione è stata la predisposizione delle misure organizzative necessarie a garantire la migliore esecuzione dell'intervento internazionale. Fra questi due opposti fattori, non vi è alcun dubbio che fosse

quella che poteva diventare la strage di un popolo si è arrestata, e i combattimenti si sono successivamente caratterizzati come scontri tra le forze in armi dei due schieramenti, forze governative e forze di opposizione. fare un macabro, lugubre calcolo delle vittime, sicuramente diremmo che dal 18 marzo in poi le vittime, se ci sono state - e ahimè ci sono state in numero inferiore rispetto a quanto era successo prima, e soprattutto rispetto a quanto sarebbe successo se fosse mancato l'intervento della comunità internazionale. Come è arrivata l'Italia all'intervento? Qualcuno ha detto che vi è arrivata troppo troppo presto, qualcuno ha lamentato che l'intervento della comunità internazionale e dell'Italia stessa sia arrivato troppo tardi. In realtà, noi riteniamo che mai come in questa occasione il Governo, confortato però, devo dirlo, dalla opinione della stragrande maggioranza della Camera e del Senato, ha scelto i tempi assolutamente adeguati alla necessità è intervenuto immediatamente sul piano umanitario, come ha ricordato il ministro Frattini. Aggiungo che il nostro è stato il Paese più impegnato nell'evacuazione di cittadini stranieri e di cittadini italiani: non ho bisogno di dirvi il numero, ma si pensi che il numero di cittadini stranieri che abbiamo evacuato è superiore di quattro volte al numero dei cittadini italiani che abbiamo evacuato. è stato il primo, come ha ricordato il Ministro, a mandare aiuti a Bengasi, ma anche a mandare aiuti alla frontiera con la Tunisia, fornendo assistenza sanitaria, trasportando e riportando a casa

alleati che ci chiedevano l'utilizzo delle basi per scopi umanitari, raccomandando, esigendo, pretendendo che ad utilizzarli fossero assetti destinati solo a scopi umanitari; perché, come ci impone la nostra Costituzione, non potevamo immaginare nessun altro tipo d'intervento senza un previo via libera, per così dire, degli organismi internazionali. Quando l'organismo internazionale, superando difficoltà insite nelle sue modalità di decisione, che prevedono come sapete la possibilità del diritto di veto, ha ottenuto della larga maggioranza dell'organo preposto alla decisione e l'astensione anche di Russia e Cina, che potevano in ipotesi porre il veto, solo in quel momento e senza indugio l'Italia si è trovata davanti alla scelta di partecipare o meno allo sforzo della comunità internazionale teso a salvaguardare, come imponeva la risoluzione, l'integrità fisica del popolo libico.

prospettare l'opportunità di un'adesione alla coalizione che si era intanto formata in esecuzione del deliberato delle Nazioni Unite al fine di proteggere la popolazione libica. Non vi era dubbio - come ci ha indicato il Parlamento attraverso il voto unanime dei presenti, con la non partecipazione al voto della che non potesse esservi scelta. Non c'è stato né entusiasmo, né ripensamento: era una scelta logica quella di offrire le nostre basi,

il nostro Presidente del Consiglio ha partecipato ad una riunione, nel corso della quale è stata presa la decisione di formare la coalizione; un documento, con il quale si decideva di agire attivamente per rendere concrete le prescrizioni la nostra adesione alla coalizione, della quale fanno parte numerosi Paesi. Se volete, ve li ricordo: Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Italia, Spagna, Canada, Danimarca, Belgio, Grecia (tutti Paesi appartenenti alla Nato), ai quali si aggiunge il Qatar.

Abbiamo messo a disposizione quattro aerei Tornado e quattro caccia F-16. Si è molto discusso

tra gli assetti messi a disposizione dall'Italia, non figurano i Tornado. Ripeto, senza contrasto: quindi non è che abbiamo negato tali assetti, ma abbiamo determinato in una cordiale

nemici. A cosa serve questo oscuramento? Si dice che questi aerei sono i primi ad arrivare in teatro e gli ultimi ad andare via, perché sono quelli che rendono possibile l'impiego di altri mezzi aerei senza che questi corrano il pericolo di essere abbattuti dalla contraerea; infatti, non appena si accendono i radar atti ad individuare gli aerei della coalizione, i nostri Tornado possono oscurarli, o semplicemente con un intervento di tipo elettromagnetico (cioè che provoca un "rumore magnetico" che impedisce ai quei radar di vedere gli aerei), o con un missile di precisione, che non ha normalmente effetti collaterali ma che insegue e distrugge l'emissione radar anche ove questa venisse accesa e immediatamente spenta, perché la memorizza, la insegue, la colpisce e l'annienta. Questi sono i mezzi che abbiamo messo a disposizione, oltre ai quattro caccia che - come è noto - hanno un compito di scorta, di accompagnamento e di messa in sicurezza. Abbiamo al di fuori della coalizione i mezzi i mezzi navali, che sono stati allertati, e rimane naturalmente in atto la copertura dello spazio aereo italiano, come avviene normalmente, normalmente, e più specificatamente in questa fase, in cui l'allerta è stata portata ad un livello più alto, in modo che quattro caccia italiani possono sempre essere in quattro caccia italiani possono sempre essere in volo in soli 15 minuti per la protezione, questa volta, del nostro spazio aereo, al di fuori della coalizione. Questo è l'apporto concreto che abbiamo dato partecipando ad una coalizione che sicuramente vede l'Italia in un ruolo - ve lo posso assicurare personalmente di grande rilievo anche politico nei confronti degli altri Paesi. Nelle riunioni che abbiamo fatto a Bruxelles, il peso e l'ascolto della nostra conoscenza delle vicende libiche è stato assolutamente notevole. I Paesi alleati sanno benissimo che non è possibile immaginare un futuro della Libia senza un ruolo politico, attivo, sociale, economico e diplomatico dell'Italia. E lo sappiamo anche noi che siamo comunque i primi a pagare le conseguenze di ciò che sta avvenendo. Lo sanno i cittadini di Trapani, che hanno visto chiuso il loro aeroporto - lo dico al senatore D'Alia e agli altri parlamentari che me ne hanno fatto domanda - sia pure solo per pochi giorni e per il tempo necessario a riaprirlo gradualmente, necessità di sicurezza. Ne stiamo pagando le conseguenze in termini di possibile pericolo di immigrazioni sempre più vaste, tra le quali bisogna distinguere quelle dei profughi da quelle possiamo definirla - immigrazione clandestina, quale quella attualmente in atto dalla Tunisia, dove non vi è guerra ma dove è venuto meno il controllo della polizia tunisina, che era presente prima dello scoppio delle vicende di cui tutti oggi siamo in grado di conoscere la portata. voglio riferire che è arrivata questa mattina al porto di Lampedusa, su richiesta del ministro degli interni onorevole Maroni, la nave italiana che ha già imbarcato 600 immigrati immigrati per trasferirli in altro luogo italiano. Certo, noi siamo consapevoli che il nostro intervento, doveroso per i motivi umanitari che abbiamo detto e per dare esecuzione alle ragioni che hanno portato la comunità internazionale

di una biblica immigrazione di profughi, che avremmo il dovere di assistere (diverso è il problema normativo riguardo l'immigrazione clandestina: parlo di profughi).

Né possiamo immaginare che l'assenza di intervento avrebbe migliorato la situazione: anzi l'avrebbe resa probabilmente ancora più drammatica, e avrebbe lasciato l'Italia più sola nella gestione ipotetica della fuga dalla Libia di migliaia e migliaia di profughi. Per questo motivo penso di poter affermare che ci siamo mossi come Governo, come Parlamento - ho l'orgoglio di dirlo almeno

Non siamo intervenuti né troppo presto, né troppo tardi. Non siamo intervenuti né con poco, né tantomeno con tanto entusiasmo: non c'è mai entusiasmo nel dover fare ricorso

Forze armate, delle quali - ve lo posso assicurare - potete tutti essere molto orgogliosi per la prontezza, l'efficienza e l'efficacia che anche questa volta hanno saputo dimostrare.

noi radicali abbiamo già espresso venerdì, nel corso del dibattito delle Commissioni riunite, la posizione per la quale vogliamo che il nostro Paese sia pienamente impegnato nell'applicazione della risoluzione n. 1973, nei suoi limiti ma anche nella sua interezza. Sicché oggi nel dibattito in corso, nei minuti che ho a disposizione, desidero soffermarmi su due aspetti che mi pare ci vedano ancora distanti, signor Ministro e signori del Governo. Il primo è la sospensione formale del Trattato. Non condivido, signor Ministro, neanche la tesi per la quale la non sospensione formale consentirebbe all'Italia, una volta passata la bufera, di avere una posizione di di maggiore preminenza nei rapporti con il nuovo Governo libico; penso esattamente il contrario. Penso che solamente un segno di discontinuità formale con il passato regime possa forse farci sperare, con il passare del tempo e con una politica diversa, di riacquisire, agli occhi del popolo libico e del nuovo Governo, quella credibilità che invece siamo andati perdendo, di errore in errore, negli ultimi anni, ma anche - a mio avviso - da prima. Per questo la risoluzione che presentiamo insiste perché il Governo assuma tutte le iniziative necessarie in base alle convenzioni internazionali per la sospensione formale del Trattato, dovuta alla violazione dell'articolo 6 del Trattato stesso da parte del Governo libico, da parte del regime di Gheddafi.

la lente della Corte penale internazionale. Il nostro Paese, che pure è stato dieci anni fa il più grande sostenitore e promotore della Corte penale internazionale, in dieci anni non ha recepito nel nostro ordinamento nazionale gli atti previsti dallo statuto della Corte. Per farla breve: se passassero da queste parti Al Bashir o Gheddafi, il nostro Paese non li potrebbe neppure arrestare. Può far piacere, ma è illegale. Dopo nove anni, anni, chiediamo al Governo un impegno, perché sappiamo bene che il disegno di legge è già uscito dai vari Ministeri ed è fermo da quel dì, forse non a caso, alla Presidenza del Consiglio.

non riesce a gestire un'emergenza di 15.000 persone, c'è da chiedersi di quale Paese stiamo parlando.

alla legalità internazionale! Di questo dobbiamo andare orgogliosi, e non di allarmismi che non si verificano neppure! Infine, signori Ministri, voglio che sia chiaro che il blocco militare serve a impedire le forniture a Gheddafi e non a bloccare

finestra") *(PD)*. Signor Presidente, signori Ministri, colleghi senatori, di fronte ad una prova così impegnativa e rischiosa come quella che stiamo vivendo a tutti chiarezza di linea politica, determinazione nel perseguirla, moderazione nell'uso della forza, legittima e necessaria,

che questa chiarezza, questa determinazione e questa responsabilità non l'abbiamo potuta cogliere nell'incredibile diserzione dal voto da parte di una forza di Governo determinante per la maggioranza; non l'abbiamo colta nel rifiuto incomprensibile del Presidente del Consiglio a venire qui oggi, analogamente a quanto fatto da tutti i leader di tutti i Paesi del mondo e in tutti i Parlamenti impegnati in questa vicenda, spiegare al Parlamento e al Paese le ragioni dell'impegno del Governo. Devo dire che non l'abbiamo trovata nel metodo, nel deludente testo e nel contenuto della risoluzione proposta dalla maggioranza. Signor Presidente, noi abbiamo cercato di fare la nostra parte. Venerdì scorso, con il nostro voto determinante, il Parlamento ha impegnato il Governo ad adottare ogni iniziativa necessaria per assicurare che l'Italia partecipi attivamente alla piena attuazione della risoluzione n. 1973 del 17 marzo 2011, ai fini della protezione dei civili e delle aree popolate sotto attacco in Libia, ivi compresa la concessione in uso di basi sul territorio nazionale. Abbiamo votato questo dispositivo in Commissione non senza preoccupazione, perché decidere l'uso, sia pur limitato e legittimo, della forza, è sempre difficile, ma lo abbiamo fatto con piena e serena convinzione. Sappiamo infatti di aver preso una decisione coerente con l'articolo 11 della nostra Costituzione, che ripudia la guerra se non per legittima difesa, ma rifiuta anche qualunque concezione neutralista o isolazionista, in favore di un impegno attivo per la creazione di un ordine mondiale giusto e pacifico. Sulla base dell'articolo 11 della Costituzione, come il Presidente della Repubblica ha ripetutamente ricordato, l'Italia non può restare indifferente rispetto alla qualità dell'ordine mondiale in termini di pace e di giustizia. Al contrario, l'Italia deve intervenire, e deve farlo attivamente, nel contesto internazionale, con il duplice vincolo stabilito dal fine, che deve essere la promozione della giustizia e della pace, e dal mezzo, che deve essere quello della legalità e del diritto internazionale come affermati attraverso la limitazione della sovranità dei singoli Stati e la promozione degli organismi multilaterali, a cominciare dalle Nazioni Unite. La costruzione di un nuovo ordine mondiale di giustizia e di pace passa oggi più che mai per il Mediterraneo, e quindi coinvolge appieno ed in prima linea il nostro Paese.

e di progresso. È nel nostro interesse nazionale aprire la possibilità di una nuova centralità del Mediterraneo attraverso una nuova stabilità, affidata non più a regimi autocratici, ma a risposte affidabili alla domanda di libertà e di democrazia dei popoli arabo-islamici. Anzi, l'unico modo per difendere e promuovere l'interesse nazionale è quello di ancorarlo ad una visione lungimirante di politica estera, che investa sulle energie di cambiamento anziché sulla conservazione di un ormai indifendibile *status quo.* *(Applausi dal Gruppo PD)*. Il nostro Governo, lo abbiamo detto più volte, a lungo si è attardato nell'illusione di poter difendere questo *status quo*, e noi abbiamo fatto il nostro dovere di opposizione, incalzando il Governo ad assumere una posizione più coraggiosa. Chi ha compreso meglio e per primo cosa si poteva muovere nel mondo arabo-islamico è stato il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, con il famoso discorso all'Università del Cairo del 4 giugno 2009. Mentre noi ricevevamo con tutti i salamelecchi del caso Gheddafi, il Presidente nero dal nome arabo, immagine vivente di una globalizzazione inclusiva e plurale, affermava la compatibilità tra Islam e democrazia, si schierava dalla parte dei popoli che si battono per il valore universale della libertà e dei diritti umani e, al tempo stesso, ripristinava il rispetto della sovranità altrui e l'opzione preferenziale per il multilateralismo, entrambi violati da Bush con l'intervento in Iraq. La dottrina del Cairo non ha evitato alla Casa Bianca esitazioni ed incertezze dinanzi al precipitare degli eventi, imprevedibile per tutti, almeno nei modi e nei tempi; tuttavia, ha consentito ed offerto un nuovo paradigma per affrontare un passaggio storico così difficile e così impegnativo come quello che riguarda il Mediterraneo. La crisi libica e l'arroccamento di Gheddafi hanno malamente complicato la situazione. Le violenze e le atrocità che Gheddafi ha commesso contro il suo popolo gli sono valse la condanna unanime della comunità internazionale, con la risoluzione n. 1970, e l'autorizzazione all'uso della forza per imporre il cessate il fuoco e proteggere le popolazioni civili, con la risoluzione n. 1973. Ora il multilateralismo deve dimostrarsi efficace sul difficile, insidioso terreno libico, costringendo Gheddafi a mollare la presa e consentendo al popolo libico di trovare la sua via verso la libertà. Noi dobbiamo essere dalla parte di questo popolo, offrire a questo popolo la sponda della legalità internazionale e dell'uso misurato e responsabile della forza. Abbiamo davanti a noi una sfida grande, signor Presidente. Cerchiamo tutti di esserne all'altezza.

Signora Presidente, signori Ministri, colleghi e senatori, la guerra civile di fatto in corso in Libia non è un fatto isolato, come sappiamo. Si inscrive in una ormai abbastanza lunga teoria di eventi importanti che segnano un distacco tra i popoli ed i regimi di molti Paesi dell'Africa settentrionale. Questo corrisponde ad una richiesta di modernizzazione, di libertà, di democrazia che si radica soprattutto nelle generazioni giovani di quei Paesi, ad alto tasso di scolarizzazione, prevalenti nella demografia di quei Paesi e che fanno sentire ancora più netto lo squilibrio che quelle dittature portano in quelle in quelle società. Questo vento di protesta si è alimentato con la circolazione delle informazioni rese possibile da Internet e dai moderni sistemi di comunicazione, e di fatto è a tutto questo che dobbiamo non soltanto la vicenda libica, ma prima di questo le vicende a cui abbiamo assistito negli ultimi tre mesi, a cominciare

pesa l'assenza di una strategia dell'Unione europea per il Mediterraneo: non ci sono più lo spirito e gli obiettivi del processo di Barcellona, paiono importanti solo le questioni migratorie di accoglienza, di cui peraltro l'Unione sembra disinteressarsi lasciando la patata bollente in mano ai Paesi di confine confine come l'Italia. Ma diciamo che sia in Italia che in Europa prevale ed è prevalsa in tutti questi anni la tendenza a preferire la stabilità dei regimi e la conservazione degli interessi economici al rispetto dei diritti umani e civili ed al sostegno dei processi di transizione democratica. democratica. La guerra in Libia si è sviluppata sotto i nostri occhi nel giro di poche settimane con la repressione sanguinosa di migliaia di civili, inaccettabile per la comunità internazionale: una situazione che ha creato gravissimi rischi per l'Italia e l'Europa dal punto di vista degli approvvigionamenti energetici, delle tensioni sull'economia, dei flussi migratori e della sicurezza dell'intera area. L'assetto futuro del Paese è estremamente incerto, ed in questo contesto dalla comunità internazionale è arrivata una dura condanna, prima con la risoluzione n. 1970 che ha deferito unanimemente Gheddafi alla Corte penale internazionale per crimini contro l'umanità, poi con la risoluzione n. ha autorizzato l'istituzione di una zona di non sorvolo con tutte le attività accessorie, sulla cui estensione evidentemente la discussione è molto aspra. La posizione dell'Italia è oggettivamente scomoda. Il trattato in sé -permettetemi di dirlo - non era una cattiva idea, al netto degli episodi folcloristici della nostra politica estera, se visto nella logica della affermazione e del riconoscimento di una responsabilità storica e del porre le basi per un nuovo rapporto di amicizia con un Paese, non con un dittatore. Questo rischia di essere l'errore. Ed è per questo motivo che vorremmo oggi che il Trattato è servito anche ad aspetti che non sono pienamente accettabili. La diminuzione - diciamo pure il crollo - degli sbarchi e dell'immigrazione è un risultato positivo, ma forse non se conseguito in questo modo, con questa sistematica violazione del diritto di asilo, di cui, secondo i giuristi, potremmo presto essere imputati noi stessi, non soltanto la Libia. Il Trattato, così com'è, è una delle cose che vorremmo vedere formalmente cadere. In questa logica, questo è uno dei punti di una risoluzione che il nuovo Polo per l'Italia ha presentato

deve andare nella logica di una condivisione degli aspetti relativi ai fenomeni migratori da parte di tutta l'Unione europea, com'è peraltro previsto dal Trattato dell'Unione europea e come era previsto dalla direttiva Kosovo del 2001. Questo è un altro dei punti che chiediamo in questa risoluzione. Le trasformazioni nel mondo arabo sono

disturbare Gheddafi" abbiamo preso timidamente le parti degli insorti, poi timidamente le parti di Gheddafi, poi l'abbiamo timidamente bombardato, però ce ne siamo detti addolorati. Io credo che forse, da adesso in poi, è bene che ci sia ben altra decisione. Siamo invece stati molto decisi con la Francia, che ha espresso una diversità politica prima ancora ancora che militare, riconoscendo gli insorti e poi inviando i caccia in tempo utile per salvare Bengasi dalla conquista da parte di Gheddafi. Soprattutto, la Francia si è resa conto che, se Gheddafi la spunta, le speranze istanze e della giovane democrazia araba sono veramente a rischio. Siamo a rischio anche noi, perché, se Gheddafi la spunta, le minacce che questo dittatore (che in passato ha fatto ricorso al terrorismo internazionale in modo sistematico) ha già formulato nei confronti dell'Italia e degli altri Paesi della coalizione sono chiare e non equivoche.

Signora Presidente, colleghi, signori Ministri, ringrazio il Governo per queste comunicazioni esaustive fornite all'Aula del Senato, che hanno messo in evidenza come l'Italia abbia fin dall'inizio, ancora prima della risoluzione dell'ONU, operato per il meglio a favore del popolo libico.

Appena l'ONU ha dato il via libera alla risoluzione n. 1973, l'Italia ha immediatamente aderito, mettendo a disposizione le basi militari e aeronautiche del nostro Paese. Ha inoltre messo a disposizione forze militari, aerei (con il compito preciso - come ha chiaramente detto il Ministro - di neutralizzare le batterie radar), Si è resa conto subito che c'era qualche piccolo problema in questo intervento rapidissimo, anche se forse tardivo rispetto ai rischi che correva Bengasi. C'era un problema di catena di comando, con un protagonismo eccessivo da parte di alcuni Paesi

Abbiamo raggiunto l'obiettivo di impedire una strage a Bengasi; è stata bloccata l'avanzata delle truppe leali al colonnello Gheddafi; ci sono ancora combattimenti complessi da evitare, in quanto si svolgono in centri abitati, dove le azioni militari dal cielo possono creare effetti collaterali. Ma abbiamo davanti il vero obiettivo: una volta raggiunto il cessate il fuoco, sarà opportuno agire in termini diplomatici e politici per fare in modo che non si assista a uno stallo dei combattimenti, che comporterebbe una suddivisione del Paese in due parti (la Tripolitania e la Cirenaica), creando quindi tutte le premesse peggiori

Signora Presidente, signori Ministri, colleghe e colleghi del Senato, la risoluzione n. 1973 ha una finalità portante e preminente, che è quella di offrire protezione alla popolazione civile della Libia, minacciata e colpita dal regime di Gheddafi. Sono preoccupanti le voci dissonanti che si levano dalla coalizione circa la linea di comando delle azioni militari, anche se i dissensi sembrano in via di composizione. Sono ancora più preoccupanti le voci dissonanti pervenute nei giorni scorsi dalla coalizione di Governo. vi è quella davvero inaccettabile che vorrebbe un blocco navale a due facce: la faccia rivolta verso la Libia, per bloccare l'approvvigionamento di materiale bellico e strategico, e quella rivolta verso l'Europa e verso l'Italia, per bloccare profughi e migranti. Se quello della protezione umanitaria delle popolazioni civili è il fine principale della coalizione, allora non è possibile ignorare alcuni elementi di fatto. Sei milioni e mezzo sono le persone che vivono in Libia, ma una parte di esse sono più vulnerabili delle altre. Più di tutti lo sono coloro che si sono sollevati contro Gheddafi. Ma vulnerabile è anche quella quarta parte della popolazione libica di altra nazionalità, costituita in parte da immigrati regolari e per due terzi da persone irregolari. Si tratta dei cittadini di altri Paesi della regione sahariana e subsahariana, la cui vulnerabilità giuridica e sociale, già evidente in tempo di pace, è destinata ad accrescersi in tempo di guerra immigrati arrivati da Nigeria, Ghana, Ciad, Mali, Somalia, Congo, Sudan, impiegati nel settore informale, oggetti di arbitrarie espulsioni, di arbitri, di violenze a sfondo razziale. Di questo universo a rischio, i più cercheranno di restare, sperando in tempi migliori; altri tenteranno di rientrare in Patria; altri ancora potrebbero avventurarsi in una traversata via mare, in cerca di un approdo europeo. L'Italia ha un interesse strategico nell'assicurarsi una posizione di rilievo tra i Paesi della coalizione, e potrebbe farlo proprio in ambito umanitario. Si pensi alla situazione paradossale degli eventuali profughi in cerca di asilo e protezione. Questi possono avanzare domanda di asilo solo se arrivano fisicamente nel Paese di destinazione (supponiamo l'Italia); ma per farlo debbono avere passaporto e visto. Altrimenti possono arrivarci solo irregolarmente, via mare, sempre che non vengano intercettati e rimandati al punto di partenza, ossia sulle spiagge libiche, cioè nel Paese dal quale fuggono. Questo è il primo paradosso. Ma esiste un secondo i Paesi europei sono vincolati dalle regole di Dublino II, secondo le quali l'esame di una richiesta di asilo compete al primo Paese comunitario nel quale la persona fa ingresso. Vengono così penalizzati i Paesi geograficamente più esposti (l'Italia per gli arrivi da Libia e Tunisia, la Grecia per gli arrivi dal Mediterraneo orientale, la Spagna per quelli dal Mediterraneo occidentale); penalizzato anche il richiedente asilo. Il cittadino tunisino che approda in Italia, ma vorrebbe andare in Francia perché lì ha parenti ed amici e potenziale lavoro, avrà la sua domanda d'asilo esaminata in Italia e qui dovrà restare se la domanda verrà accolta. Ed ecco una proposta. Invece di invocare una barriera protettiva navale che impedisca il passaggio alle persone in fuga, l'Italia ponga a disposizione della coalizione mezzi, risorse e competenze e richieda preminenza nella gestione delle operazioni di protezione per le popolazioni migranti. Proponga, con l'accordo della UNHCR, dell'Unione europea, dei Paesi della coalizione, delle eventuali autorità provvisorie libiche, di Tunisia ed Egitto la costituzione di presìdi attrezzati e con buone risorse, da situarsi in zone protette nel territorio libico e nei Paesi confinanti, nelle quali i profughi vengano posti sotto protezione internazionale e le loro domande

(gran parte dei richiedenti avrebbero potuto intraprendere una traversata verso l'Italia). Una proposta consimile, consigliata e giustificata dall'emergenza, potrebbe poi tradursi nel pilastro di un nuovo assetto delle politiche migratorie nel Mediterraneo. Non è forse questo quel che chiede l'Italia? E come potrebbero essere contrari i leghisti? Ma ci sono altri vantaggi. Il primo è umanitario ed è inerente il fatto che, dal 2002 a oggi, 4.000 migranti sono morti nelle traversate del canale di Sicilia: la necessità di intraprendere rischiose traversate si ridurrebbe ed altre stragi sarebbero evitate. Il secondo è politico internazionale: ci distingueremmo ad occhi africani per un'azione umanitaria di alto profilo e non solo per la partecipazione ad operazioni belliche. Il terzo vantaggio è invece politico-europeo, poiché porremmo basi concrete per la revisione del regolamento Dublino II, invocata da anni presso partner europei duri d'orecchio, ma anche resi scettici da un atteggiamento italiano che nelle questioni migratorie più Europa quando fa comodo e meno Europa quando le regole che essa esprime ci mettono in imbarazzo. Signori

la sua posizione ha avuto un grandissimo merito: dapprima ha portato un clima di conciliazione (poche volte su questioni di questa natura si è trovata una convergenza

ha dato una propria interpretazione (la Francia, forse, è stata la più intraprendente). Ma se un incidente provocato dall'intraprendenza francese avesse creato una situazione oggettivamente difficile, chi avrebbe dovuto rispondere? Probabilmente tutti, e l'Italia

sull'Algeria e sulla Costa d'Avorio sta, probabilmente, cercando un altro magazzino africano da cui rifornirsi. Ma anche questo sarebbe scadere in discussioni

perché i rifugiati non sarebbero stati sopportabili esclusivamente dall'Italia. Anche a questa domanda è venuta una risposta: il Consiglio affari esteri dell'Unione europea, infatti, proprio lunedì ha stabilito ed affermato il principio di solidarietà nei confronti degli Stati membri che sarebbero stati più direttamente interessati dai movimenti migratori. quella che all'inizio era una posizione di strappo della Lega nei confronti del Governo è divenuta poi la posizione del Governo e del Paese, ed oggi è divenuta anche la posizione di tutta la coalizione, al punto che anche la Francia aderisce a questa linea.

Per assurdo, i repubblicani sono stati meno aspri nel criticare il Presidente, e perfino il *Tea Party* ha liquidato la vicenda, sostenendo che la Libia non rappresenta una minaccia per gli Stati Uniti d'America. Stranamente abbiamo trovato una posizione estremamente ragionevole da parte della Turchia, altro Stato che inizialmente era assai contrario all'intervento, mentre

Gheddafi chiede. L'interesse nostro è che la situazione non segua questa direzione in quanto, ahimè, disagi e disastri successivi non vorremmo nemmeno immaginarli.

altrettanto difficile è pensare di mantenere al potere chi ha attaccato militarmente i propri oppositori ed ucciso senza pietà la propria gente che protestava.

ad esempio quelle che saranno impossibilitate ad onorare i contratti in essere, che fossero assicurate nei pagamenti e precluse da eventuali azioni legali per inadempimenti contrattuali. pregiudicato il nostro approvvigionamento energetico al punto da dover riattivare gli accordi bilaterali, sempre in materia energetica. Infine,

il Governo di un Paese che scopre con sei mesi di ritardo che ha ospitato con tutti gli onori, rischiando perfino di riceverlo in quest'Aula, un dittatore deferito alla Corte penale internazionale o ha cattivi Servizi di informazione oppure ha una politica estera fallimentare. Il Governo di uno Stato che ispeziona, ma non spara, in un Paese con cui ha stretto un patto anche militare scoprendo (se lo avete scoperto) di avere venduto armi da guerra per milioni di euro a chi le usa contro i propri cittadini, ha una politica di difesa ed una politica estera fallimentari. Il Governo di un Paese che non rispetta le convenzioni sul *non-refoulement* e non ratifica le direttive dell'Unione europea sul rimpatrio volontario, e poi chiede aiuto alla stessa UE in maniera un po' furbesca, e manca del suo Ministro degli affari europei ha una politica europea fallimentare. Le rivoluzioni popolari nate in Tunisia, in Egitto e in Libia, ma che non si fermano lì, perché sono anche in Bahrein, nello Yemen, e perfino in Arabia Saudita, chiedono un Paese che colga il nesso tra popolo e democrazia che si sta sviluppando in Paesi dove tradizionalmente si era ritenuto impossibile coniugare aspirazioni nazionali e sociali e democrazia. Non solo: la democrazia invocata dalle piazze africane ed arabe ha allontanato lo spettro dello scontro di civiltà e della "fine della storia". Per questo, noi dobbiamo sostenerla. Dovremmo sentire il grido di libertà che ci giunge da quelle piazze e predisporci a politiche organizzate di accoglienza ed asilo politico, di flussi immigratori in un quadro europeo, di cooperazione allo sviluppo e di fraternità (altro che solidarietà!). Gli Gli articoli 10 ed 11 della nostra Costituzione ce lo impongono; la nostra appartenenza alle Nazioni Unite ce lo impone; il nostro interesse nazionale ce lo consiglierebbe. Tuttavia, il vostro Governo festeggia il centocinquantenario d'Italia come il "re tentenna": voi tentennate, trattate, balbettate, lisciate il pelo all'autocrate trionfante e bastonate lo stesso solo quando è nella polvere. La demagogia non basta più: senza l'ONU e l'Unione europea saremmo ormai declassati come Paese nel mondo. Se non fosse tragico, sarebbe comico constatare come accanto all'operazione "Alba dell'Odissea" sia in atto nel nostro Paese con il Governo Berlusconi la missione "A luci spente sul viale del tramonto".

credo di essere quel senatore cui lei si è rivolto e che invece ha chiamato senatore D'Alia, al quale certamente mi legano profondi rapporti di amicizia e di stima, ma ritengo che nella fattispecie vi sia stata una certa confusione. Intervengo per una questione certamente di dettaglio, non di alto e nobile profilo di politica internazionale, ma di concreto dramma del territorio.

si è concentrato l'utilizzo sulla base di Trapani Birgi e si è disposta l'immediata chiusura del terzo scalo della Sicilia, che veicola circa 2 milioni di passeggeri

che potevo dire oggi nel corso del dibattito su una delle mozioni da me presentate e che immagino la Presidenza, e penso anche il Governo, abbiano ritenuto che, essendo questione *de minimis*,

credo che il Governo italiano abbia interesse a ridurre al minimo le conseguenze negative in danno di singole porzioni del territorio nazionale causate da attività collegate a operazioni militari. Volevo segnalarle che questo così non è per la provincia di Trapani, che con i suoi due milioni di passeggeri veicolati dall'aeroporto di Trapani Birgi ha segnato un 53 per cento in più di presenze straniere, unica Provincia in controtendenza in Italia nell'afflusso turistico,

su sette basi messe a disposizione dal Governo italiano, oggi Trapani sia descritta come uno scenario di guerra su tutte le televisioni italiane. Credo che questa sia una questione importante non solamente dal punto di vista del dettaglio, cui certamente lei potrà riferirsi: perché l'Italia ha la necessità di concentrare su una sola base la stragrande maggioranza delle sue attività? Forse perché le altre basi non sono in grado di attivarsi, e quindi c'è bisogno di sopperire? di sopperire? Questo è molto preoccupante sul panorama strategico nazionale. Noi siamo in questo momento vittime, anche dal punto di vista mediatico, di una rappresentazione che ci fa apparire quasi in zona di guerra, e questo non può essere per il territorio trapanese, e non può essere per il territorio siciliano. Bisogna differenziare le presenze, perché si dia la sensazione di un equilibrato riparto dello sforzo e quindi anche del supporto.

Non so se di questo lei è al corrente; certamente non sono stati messi al corrente della chiusura dell'aeroporto civile di Birgi, per loro stessa ammissione, il Presidente del Consiglio, il Ministro dei trasporti, i ministri siciliani Alfano e Prestigiacomo, che sono prontamente intervenuti ma, ahimè, in questo momento senza esito. Il protrarsi di soli pochi giorni di quella chiusura creerà alla Sicilia un danno superiore alla chiusura di Termini Imerese, perché non è un problema di concentrazione dell'occupazione, ma di diffusione dell'occupazione, che noi abbiamo costruito con anni di durissimo lavoro, con risorse, cari colleghi della Lega, tutte del territorio, che hanno portato ad una esplosione dell'aspetto turistico. Il nostro petrolio lo avevamo e lo abbiamo a casa e non è quello che bisogna andare a conquistarsi con i carri armati. *(CN)*. Signora Presidente, onorevoli senatori, signori Ministri, l'intervento aereo della coalizione dei volenterosi, attuato sulla base della risoluzione dell'ONU n. ha impedito alle forze lealiste la conquista di Bengasi e di fatto la sconfitta per il movimento degli insorti. Attualmente la *no fly zone* è stata implementata e le difese antiaeree libiche disabilitate, ma la situazione appare ancora di stallo. I ribelli controllano una parte della Cirenaica ed alcune province assediate della Tripolitania, come Misurata o Zenten; le forze di Gheddafi controllano il resto del Paese. Dopo l'avvio dei *raid* gli insorti hanno cercato di riprendere il controllo di Al Adabiya, in Cirenaica, ma sono stati respinti dalle forze lealiste asserragliate nella città stessa. In tale contesto, l'utilizzo degli attacchi aerei per la protezione dei civili, come previsto dalla risoluzione dell'ONU, è appunto inibito dal fatto che le forze di Gheddafi operano all'interno delle città, dunque ci sono alte probabilità di provocare gravi danni collaterali che tutti noi ben possiamo immaginare. Sul piano politico-diplomatico la comunità internazionale sta nel frattempo discutendo di un passaggio del comando dell'operazione, cioè dalla coalizione dei volenterosi alla NATO. A tal proposito, un primo accordo è stato trovato tra il presidente Obama, il primo ministro britannico Cameron e il presidente francese Sarkozy, anche se la Francia vorrebbe limitare il comando NATO alle questioni operativo-militari, continuando a chiedere una cabina di regia politica, cioè esterna al Consiglio Nord Atlantico, cosiddetto NAC. Allo stesso tempo, in sede ONU, la Russia sta premendo per una propria mediazione che porti alla stipula di un cessate il fuoco tra le due parti in conflitto. L'andamento degli scontri sul campo sembra del resto andare in questa direzione, con le due parti impegnate a garantirsi il controllo della più ampia fetta di territorio possibile in vista di uno stop delle operazioni militari. In tal caso, la Libia si dividerebbe in due unità: Tripolitania, Fezzan e Golfo della Sirte fino a Brega da una parte, e Cirenaica dall'altra. Questo scenario potrebbe essere favorito anche dal fatto che il regime di Gheddafi è tutt'altro che isolato sul piano internazionale. Il colonnello, infatti, confida nelle divisioni tra i Paesi occidentali e gode ancora di importanti entrature nel mondo arabo e islamico, in importanti Paesi come l'Algeria o la Siria o lo stesso Pakistan o nei Paesi dell'Europa dell'Est, dalla Bielorussia fino all'Ucraina. A tutto ciò bisogna aggiungere la sfera di influenza, costituita in oltre venti anni di attività, di cui può disporre in tutto il Sahel, e che costituisce fonte di supporto politico, soprattutto presso alcuni Governi come quelli del Mali, del Ciad e del Niger, Paesi che potenzialmente costituiscono un bacino di reclutamento di miliziani e mercenari praticamente inesauribile. È necessario dunque accelerare una risoluzione politica della crisi, tenendo ben presente che la protezione e la sicurezza della popolazione civile è lo scopo per il quale l'ONU ha autorizzato gli Stati membri e, nella fattispecie, quelli che abbiamo definito coalizione dei volenterosi, a intraprendere tutte le misure necessarie affinché questo Signora Presidente, la missione in Libia è stata decisa tardi ed è cominciata male, ma è interesse di tutto il Paese che riesca.

il possibile per fermare i massacri dei civili: ricordiamolo, perché dall'intervento odierno di qualcuno sembra trapelare che il conflitto e la violenza siano cominciati dopo l'intervento. Ricordiamo le immagini delle fosse comuni sulle spiagge,

Oggi il Partito Democratico conferma con serietà, senso di responsabilità e senza furbizia e ambiguità la posizione di voto che ha espresso in Commissione, che riconosceva nella risoluzione ONU quello che oggi deve fare la comunità internazionale, nello stesso spirito di quella mirabile sintesi che il presidente Napolitano ha fatto dicendo che cosa è necessario fare. Egli ha ricordato che un Paese come il nostro e un continente come l'Europa non possano essere sordi alle richieste di democrazia e libertà che salgono dai popoli del risorgimento arabo. Il capitolo 7 della Carta delle Nazioni Unite, così come la nostra Costituzione, autorizza l'uso della forza per evitare tragedie umanitarie; non un uso della forza, quindi, a fini di sopraffazione, ma per mettere fine ad una sopraffazione. È per questo che si è mossa l'azione militare. siamo anche soddisfatti che oggi ci sia un coordinamento del comando all'interno della Nato, perché la confusione rispetto alla catena di comando proprio quando c'è un'azione militare è il peggio che si possa fare: è assolutamente deleterio. Fa male a tutti noi sentire rombare i motori dei caccia, vedere il fumo delle bombe sganciate. Quindi, c'è della sofferenza nell'assumere queste decisioni, e sarebbe sbagliato non sottolinearlo. Ma è un assenso che comunque diamo con determinazione, senza tentennamenti; quindi con sofferenza, ma senza incertezze, perché la mancanza di chiarezza in decisioni di questo tipo può essere causa di sofferenze maggiori. Dispiace, quindi, che nella risoluzione della maggioranza non si sia riproposto il dispositivo asciutto e netto che abbiamo votato in Commissione. Ci appare un testo confuso, che sembra più il frutto di una mediazione utile per tenere unita una maggioranza che sembrava deragliare rispetto al mandato richiesto dalla risoluzione dell'ONU; una maggioranza che - non possiamo non dirlo negli ultimi giorni ha dato segni di deviazione, quando invece serviva la massima compattezza. Una linea composta che peraltro, invece, abbiamo ritrovato oggi nelle relazioni dei due Ministri. come ha detto il senatore Tonini, è una sfida alta e bisogna esserne all'altezza. Ci dispiace che oggi, almeno nei testi che ha presentato oggi la maggioranza, quella compattezza che abbiamo ritrovato in Commissione non potrà essere ricomposta.

una zona di non possibilità di sorvolo, la mitica *no fly zone,* che è entrata da qualche settimana nel nostro lessico abituale, non può mai essere la gentile concessione di un altro Paese. Per instaurarla e per farla rispettare c'è da abbattere dei caccia, da distruggere batterie antiaeree, da rendere inutilizzabili dei radar, e via dicendo. Sicché, rispetto a venerdì pomeriggio, quando, con molta puntualità e con molta onestà intellettuale, sulla base delle informazioni di cui disponevano, i ministri Frattini e La Russa ci hanno informato sulle misure, sugli ambiti, sui limiti, sulle implicazioni della (evidentemente allora un problema di coordinamento, di una meno disordinata catena di controllo e di comando non si poneva ancora) tutto è stato immediato. Dopo le giornate di sabato e di domenica, abbiamo avuto una sguaiata e sgradevole impressione. Ci è sembrato che a loro modo i francesi volessero una guerra affidata soltanto ai generali, il che non è un'ipotesi di scuola, ma piuttosto un incubo, quando si verifica. Invece devo dire che dalla giornata di lunedì l'aver identificato l'idea di un coordinamento della NATO serve ad assicurare un profilo politico (non tecnico, amici francesi) all'intervento occidentale. Appartengo ad una generazione di democratici italiani per i quali la NATO non è mai stata un riferimento tecnico, ma sempre un riferimento politico, anzi etico- politico, potrebbe dirsi. dirsi. Fino a ieri sembrava allora francamente inspiegabile come la Francia di Sarkozy sulla Libia potesse nutrire la stessa avversione all'atlantismo e agli Stati Uniti con cui la Francia di Chirac e de Villepin ai tempi dell'Iraq aveva gratificato, in sede di Nazioni Unite e non solo, l'azione della diplomazia e della politica internazionale. Quindi, credo toccasse all'Italia (e bene ha fatto nelle ultime 36 ore il Governo italiano a farsene interprete), proprio in quanto Paese amico degli Stati Uniti, della Francia e anche della Germania, nonché Paese attento alle connessioni europee del proprio ruolo politico far valere, senza ipocrisie, l'opportunità di un comando NATO. Questo vale guardando la Libia, sia da Bengasi che da Tripoli. Ha detto bene il ministro Frattini: non possiamo scontare una divisione geopolitica. Ecco perché ho apprezzato la sobrietà del Governo nel renderci informati, ma non informatissimi, di quello che si sa di Bengasi. Francamente, la contrapposizione fra gli amici di Bengasi - tutti e soltanto idealisti dei *droits de l'homme* francesi - e quelli attenti a Tripoli - tutti e soltanto vedovi dell'affarismo gheddafiano è sbagliata, superficiale e cinica, ed è triste che si sia riprodotta in quest'Aula un'eco di tal genere. Lo dice uno che, fruendo delle condizioni di libertà dei provvedimenti *bipartisan*, votò contro il fatidico accordo un'ultimissima considerazione, signor Ministro. È giusto aprire il discorso anche in questi giorni, fin da adesso, ad una solidarietà europea con i Paesi più esposti a ricadute in in termini di sfollati (15.000 sfollati). Ha fatto bene il ministro La Russa, l'altra sera, ad aver un moto di solidarietà con la cittadinanza e con l'amministrazione di Lampedusa. Guardate che Lampedusa trasformata in una latrina a cielo aperto è una tragedia dell'Italia e dell'Europa, ed è cinico che in sede di Conferenza Stato-Regioni si siano sentiti gli egoismi delle Regioni più forti.

da una strategia del Governo di barriera protettiva navale degli sfollati. Di questo non ha parlato nessuno, ed è disonesto attribuire al Governo un'intenzione che non ha per polemizzare contro qualcosa di astratto.

innanzitutto intendo esprimere la preoccupazione, la forte preoccupazione - mia personale e dei colleghi del Gruppo dell'Italia dei Valori - per i gravi eventi che si stanno verificando in Libia. Vorrei anche rappresentare la vicinanza alla popolazione italiana e in particolare a quella di Lampedusa, fortemente preoccupata per il crescente numero di immigrati in arrivo sulle nostre coste dai Paesi del Nord Africa. Colleghi, non posso però non sottolineare l'assenza del presidente Berlusconi. Nemmeno fossimo in tribunale! È una vergogna. Non solo non si presenta a rispondere ai giudici riguardo ai processi in cui è coinvolto, ma ora addirittura scappa vergognosamente e irresponsabilmente anche di fronte ai suoi doveri istituzionali.

È vergognoso, ma è ovvio: maggioranza e Governo non sono ancora riusciti a scegliere una linea comune. È una miseria. Non dovrebbe essere, invece, per il Presidente del Consiglio un bisogno impellente quello di riferire davanti al Parlamento? Non ve lo chiedete anche voi, colleghi del centrodestra? La situazione in Libia, purtroppo, è sempre più grave. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 1973 ha autorizzato l'applicazione di una *no fly zone* sulla Libia e ha acconsentito che siano messi in campo tutti i mezzi necessari per proteggere i civili dalle forze del *leader* libico Muammar Gheddafi. Il 18 marzo scorso le Commissioni esteri e difesa di Camera e Senato hanno approvato una risoluzione che dà mandato al Governo ad agire in base ad una risoluzione dell'ONU sulla Libia; così è scattata l'operazione Odissea all'alba, cui partecipano al momento Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada e, frettolosamente Italia. Sono ormai diverse centinaia i missili lanciati sugli obiettivi cosiddetti sensibili del colonnello Gheddafi. L'Italia, se è vero che all'inizio non ha preso parte attivamente ai *raid* limitandosi a fornire un importante supporto logistico attraverso la messa a disposizione di ben sette basi militari, negli ultimi giorni ha fatto alzare in volo anche i propri aerei per realizzare missioni di attacco sul suolo libico. Si tratta di un supporto che mette il nostro Paese di fronte a gravi e possibili ritorsioni del regime di Gheddafi. ancora una volta mi trovo a ricordarle che, in base alla nostra Carta costituzionale, in questo Governo lei è Ministro della difesa, non altro. Spero abbia capito a cosa mi riferisco. Eppure ormai in Italia non si contano più i bombardieri e gli intercettori che decollano dalle nostre basi. È importante rispettare la risoluzione dell'ONU abbiamo sottoscritto - ma Gheddafi si sente fortemente tradito dal vostro Presidente del Consiglio. «Berlusconi - ha detto Gheddafi - era un amico» «Era il mio "bacia-mano"» ha tenuto a specificare. Il dittatore, solo poche ore fa, ha parlato dalla sua residenza dichiarando che il complotto fascista, così ha definito l'intervento ONU, finirà nel cestino della polvere della storia. Non dimentichiamo che il collasso del regime del colonnello Gheddafi potrebbe avere per il nostro Paese importanti riflessi. La Libia è il nostro primo fornitore di petrolio e il quarto di gas; gli investitori libici sono attivi in diversi settori strategici della nostra economia. Ricordiamo tutti benissimo che l'Italia, oltre ad aver firmato il Trattato d'amicizia, che l'Italia dei Valori e qualche altro piccolo partito non hanno votato, convintamente (e questi sono i risultati) si è impegnata a versare alla Libia una tangente di cinque miliardi di dollari, formalmente a titolo di risarcimento per le efferatezze del nostro colonialismo, ma di fatto pagamento per il controllo dei flussi migratori: un ricatto al quale il vostro Presidente del Consiglio ha deciso di sottostare. L'Italia dei Valori, tra le richieste avanzate con la sua risoluzione, ha anche chiesto che il Governo si impegni a prevedere velocemente la sospensione immediata del Trattato d'amicizia del febbraio 2010. Per l'Italia e non solo è una situazione di grande allerta. Occorre muoversi con fermezza. Occorre che tutti i Paesi rispettino la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU e che il Governo e la maggioranza si impegnino con serietà a fronteggiare questa grave emergenza invece di pensare ai propri interessi: è disonorevole che non riescano a trovare una linea comune fuori dalle logiche di partito. Occorre scongiurare il rischio che alcune Nazioni vadano oltre il mandato delle Nazioni Unite per fini nazionalistici differenti da quelli umanitari. Non sono così certo, infatti che tutte le Nazioni si siano buttate a capofitto contro Gheddafi solo perché lo giudicano un uomo abbietto, solo perché mosse dal desiderio di scongiurare gli attacchi e le violenze contro il popolo libico. Diciamolo, in queste gravi situazioni, è facile avere paura di dire le cose come stanno. A nome del Gruppo dell'Italia dei Valori, sono a chiedervi, signori Ministri, in rappresentanza di una persona che doveva essere qui come Presidente del Consiglio, oggi latitante nella sua Aula, che il Governo si impegni a dare seguito a quanto disposto in sede ONU con la risoluzione n. 1973, anche vigilando affinché siano rispettati i limiti di mandato. Sarebbe doveroso che il Governo provvedesse continuamente e tempestivamente a tenere informato il Parlamento sulla situazione libica. Sarebbe opportuno che il Presidente del Consiglio - lo ripeto, quello che non c'è mai non si tirasse indietro anche di fronte a questo impegno, che è istituzionale ed importante, e sappiamo bene che per gli impegni seri e istituzionali il Presidente è sempre pronto a latitare e a non essere presente. Sarebbe altrettanto doveroso che l'attuazione stretta e rigorosa della risoluzione ONU n. 1973 avvenisse nel pieno rispetto dell'articolo 11 della Costituzione. Ricordo, come ho già fatto in altre occasioni, al ministro La Russa, sempre senza polemica, che la nostra Carta fondamentale recita: «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali». Comincerò da oggi a regalare al ministro La Russa un libricino della Costituzione, ogni giorno, evidenziando l'articolo 11, che a volte dimentica. Signor Ministro, speriamo che almeno questa volta gli enunciati della nostra Costituzione non rimangano solo parole. Come tutti sappiamo, inoltre, la crisi in questa parte del Mediterraneo sta provocando, e continuerà a provocare, una crescita degli sbarchi verso le nostre coste, corridoio storico per l'accesso e il transito verso l'Europa. Proprio per questo, nella nostra risoluzione abbiamo scritto vogliamo chiedere all'Unione europea e ai singoli Stati membri, oltre al supporto economico, di farsi anche carico dell'accoglienza degli immigrati, del loro soccorso in mare, nonché del successivo smistamento.

del problema Lampedusa e del problema immigrati, e non solo del problema delle basi, per fini esterni, poi. Dobbiamo risolvere i problemi interni. Questa è la parola che non riuscite ancora a capire

L'Europa è parsa da subito refrattaria e reticente, se non a tratti addirittura indifferente al problema. In verità il Governo italiano non ha esercitato alcuna pressione sul problema degli immigrati, ma si è solo preoccupato di dire sì alla destinazione d'uso delle basi aeree in Italia, tralasciando la problematica dei flussi migratori, facendo così esplodere il caso Lampedusa e destinando alle televisioni di tutto il mondo l'immagine del Governo italiano come incapace a risolvere ancora una volta i problemi interni. Tutto, con l'unico risultato che la Francia e l'Inghilterra possono così avere la possibilità di entrare

ha chiesto che il Governo si impegni a predisporre piani di intervento più efficaci, più forti, più seri, richiedendo all'Unione europea ed ai singoli Stati membri, oltre al supporto economico (che, è vero, è molto importante, ma non basta), anche e soprattutto di farsi carico dell'accoglienza degli immigrati, del loro soccorso in mare e del successivo smistamento, nonché a valutare l'opportunità di promuovere e sostenere fattivamente proposte di modifica della normativa vigente in materia di immigrazione. Noi dell'Italia dei Valori ripetiamo che così non basta, che occorre fare di più in relazione alla problematica degli ingenti flussi migratori in corso. Signor Ministro della difesa, signor Ministro degli affari

Abbiamo elencato alcuni punti, e tra questi vogliamo evidenziarne uno credo sia importante per farvi riflettere: l'Italia deve appoggiare con forza anche l'adozione dei provvedimenti di giustizia internazionale, per fornire prove decisive e inoppugnabili dei crimini commessi dal dittatore dittatore Gheddafi. Vorrei concludere perciò con una frase di Padre Wresinski, sacerdote ormai scomparso, da sempre dedito alla tutela dei diritti dei diritti umani:«Laddove gli uomini sono condannati a vivere nella miseria, i diritti dell'uomo sono violati. Unirsi per farli rispettare è un dovere sacro». Mi auguro che questo possa essere di stimolo e d'insegnamento a voi. Signora Presidente, intervengo per illustrare la risoluzione unitaria presentata dai senatori dell'UDC, dell'ApI, di FLI, dello MPA e dei Repubblicani. Il Mediterraneo, signor Ministro, a dispetto anche di una indifferenza più o meno lampante dell'Europa, torna a recitare oggi un ruolo di primo piano, seppure in uno scenario di guerra e di rivoluzione. Fernand Braudel, storico che tutti ricordiamo, ha sempre sostenuto la centralità politica, economica e culturale del Mediterraneo che oggi torna alla ribalta per la fine dei regimi che per troppi anni hanno oppresso le popolazioni arabe. Ciò che è apparso chiaro a tutti è che è che le migliaia di giovani non organizzati dall'esterno che si sono ritrovati nella volontà di lottare per la libertà, la dignità umana, la democrazia e la Costituzione hanno espresso un'aspirazione incomprimibile per la quale sono disposti a tutto. L'Occidente, dal canto suo, ha salutato certo positivamente queste insurrezioni dell'Egitto, della Tunisia e di altri Stati. È iniziato così - si è detto - il riscatto del mondo arabo dall'oppressione dei regimi autoritari e corrotti che avrà i suoi tempi e le sue difficoltà, ma che va rispettato, aiutato diplomaticamente, così come lei ha sostenuto nella relazione che ci ha fatto, anche perché non si fermerà. Ciò che sta accadendo in Libia è però diverso da ciò che è accaduto negli altri Paesi nordafricani. L'insurrezione della Cirenaica fa riferimento ad antiche fratture all'interno della stessa società libica ed è rivolta prevalentemente contro Gheddafi e contro la sua tribù. Conosciamo poco del Consiglio rivoluzionario di Bengasi, che la Francia, con una mossa repentina, aveva già quasi riconosciuto quando invece dovrebbe essere riconosciuto da tutti i Paesi che partecipano all'operazione, facendo peraltro capire di essere pronta ad agire anche da sola. Il protagonismo di Sarkozy ci ha lasciato interdetti; ha motivazioni che possono essere giustificate e giustificabili, ma che certamente non riguardano il problema centrale di tale questione. Lui ha spinto fortemente, come Capo di Stato francese, perché si addivenisse alle risoluzioni che l'ONU ha poi pronunciato, coinvolgendo lo stesso Presidente degli Stati Uniti, che non poteva tirarsi indietro per gli interessi politici ed economici ingenti che ha in Oriente e nei Paesi del Nordafrica. Molti Stati si sono allineati, mentre altri, come la Germania, la Cina e la Russia, si sono defilati. Poi tutto è precipitato di fronte alla determinazione di Gheddafi di soffocare nel sangue la rivolta e di procedere ad una repressione violenta contro il suo stesso popolo, ingaggiando financo mercenari, tanto che la stessa comunità internazionale ha pronunciato una decisiva condanna nei confronti dello stesso Gheddafi. Di fronte a tutto questo, l'ONU ha votato due risoluzioni, la n. 1970 e la n. che hanno messo a fuoco la determinazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sottolineando l'esigenza di addivenire ad una soluzione della crisi e di dare risposta soprattutto alle legittime esigenze del popolo libico. A tal fine, si sono sottolineate anche le normative sui diritti umani e sui profughi, normative internazionali che vanno rispettate. Gli Stati membri sono stati autorizzati a prendere tutte le misure per proteggere la popolazione civile. La stessa rivolta di cui abbiamo parlato, che si è scatenata soprattutto nella Cirenaica e che sembra in qualche modo essere stata sobillata dai servizi segreti occidentali o da Paesi che hanno tanto da guadagnare da questa guerra e dal rovesciamento del regime di Gheddafi, si è però configurata in una maniera tale che non possiamo permetterci di ignorarla in nessun modo: dobbiamo dare esecuzione a quanto stabilito dalla risoluzione delle Nazioni Unite. Si dice che nessuno se l'aspettava, signor ministro Frattini, ma ancora una volta il gioco dell'ipocrisia a mio avviso tiene banco. È come se la disinvoltura con cui il nostro Presidente del Consiglio ha trattato la politica estera non abbia sollecitato riflessioni serie sia in chi gestisce la politica estera americana sia in chi la gestisce a livello europeo, soprattutto a livello francese. Personalmente giudico legittimo e positivo per gli interessi dell'Italia, non solo in campo energetico, ma anche per ciò che riguarda il controllo dei flussi migratori, gli impegni con le nostre banche, con l'ENI e con le nostre grandi imprese. Esso ha coronato peraltro gli sforzi già compiuti dai precedenti Governi di centrosinistra,

ci ha in qualche modo frenato; questo non può essere disconosciuto. Anzi, signor Ministro, è sembrato paralizzare lo stesso Governo e il Presidente del Consiglio in uno stato confusionale e contraddittorio, contrabbandato poi con il principio della prudenza e con quello della Al contrario, noi pensiamo invece che la vicenda della Libia ci chiamasse e ci chiami ad un ruolo primario, per la storia passata e per la storia presente che ci accomunano, oltre che per la vicinanza geografica. Il futuro di una Libia liberata dalla dittatura ci riguarda più di altri e richiede il concorso attivo di tutto il nostro Paese.

La voce dell'Italia si è finalmente fatta sentire a livello della Comunità europea tramite la sua persona, signor ministro Frattini. Lei ha chiesto che il comando della missione passi alla NATO, e noi siamo d'accordo, offre maggiori garanzie e dispone di mezzi tecnici e organizzativi all'altezza di una situazione così delicata e difficile. Il Presidente del Consiglio ha chiesto anche una più chiara definizione degli obiettivi della missione, che non sembra contemplare, quanto meno non in maniera precisa e chiara, la destituzione di Gheddafi, ma semplicemente la *no* *fly* *zone*, l'embargo e la protezione dei civili, alla quale siamo tutti tenuti, Italia in testa. Naturalmente la *no* *fly* *zone* a nostro avviso richiederà un grande numero di mezzi e di *intelligence,* per cui è chiaro che non si può pensare ad un comando tripartito, ma va pensato, e con urgenza, un comando unificato sotto la NATO e sotto il suo ombrello protettivo, dentro il quale

situazione che dobbiamo affrontare. Tuttavia, se non ci sarà un'iniziativa politica coerente e unitaria, difficilmente potremo raggiungere questi obiettivi, che desideriamo e che abbiamo saputo evidenziare con queste risoluzioni. Bisogna uscire dall'atmosfera dei veti incrociati. Non si possono sottolineare sempre righe e righine: occorre secondo noi una massima convergenza e un'unità nazionale a sostegno anche delle Forze armate e dell'iniziativa che il nostro Paese, seppur lentamente e con gravi difficoltà, ha cominciato ad intraprendere a testa alta.

Chiediamo che l'Italia partecipi attivamente...

a proporsi come capofila di un grande piano euro-atlantico di rilancio della cooperazione mediterranea e ad intervenire nei confronti dell'Unione europea perché si possa soddisfare una politica

in vista della trasformazione della stessa da organo di puro coordinamento degli interventi, qual è oggi, a organo di gestione delle crisi legate anche ai fenomeni migratori e, in particolare, alla costituzione di una reale politica nazionale dell'immigrazione, mai avviata in Italia al contrario di tutti gli altri Paesi europei. generale; a favorire la tempestiva approvazione dei disegni di legge pendenti in Parlamento di adeguamento della normativa interna allo Statuto della Corte Penale Internazionale ai fin di colmare una grave lacuna del nostro ordinamento;

c'è stato un solo voto contrario. Escludendo in modo esplicito l'impiego eventuale di una forza di occupazione straniera sul territorio libico, la risoluzione ha inteso raggiungere l'immediata cessazione del fuoco e l'immediata fine degli attacchi contro la popolazione inerme. In sintesi,

piedi di una repressione feroce. Tutto quello che poi è seguito dal 17 marzo ad oggi ha dimostrato, purtroppo, una grande divaricazione tra le ragioni della cosiddetta *Realpolitik* e le ragioni morali e politiche di un completo e disinteressato sostegno verso il popolo arabo. Sul quotidiano dei

ultima roccaforte degli insorti, cadesse nelle mani del *rais*, saremmo posti di fronte non solo alla sconfitta di coloro che in Libia chiedono libertà e democrazia, ma a una tragica battuta d'arresto per tutti quei movimenti che hanno dato vita alla primavera del mondo arabo». Molti Paesi occidentali - e non soltanto l'Italia - si trovano oggi a fronteggiare un'imbarazzante situazione di palese incoerenza: da un lato, la *Realpolitik* che induce a trattare con chiunque, pur di garantirsi le materie prime (in questo caso il petrolio); dall'altro lato, il diritto-dovere di intervenire in Libia a difesa della democrazia e della libertà. Accantonando temporaneamente i risvolti politici, sono evidentemente i problemi economici quelli che poi prendono il sopravvento. Il prezzo del petrolio ha superato ieri l'altro i 114 dollari al barile gettando una seria ipoteca sullo sviluppo di molti Paesi, a cominciare dall'Italia. Tuttavia, quando termineranno le operazioni militari si apriranno nuovi scenari. Per l'amministratore delegato dell'ENI è prevedibile che chiunque è al potere in Libia avrà bisogno di estrarre petrolio per superare l'attuale fase bellica e per iniziare la ricostruzione. Detto questo gli esperti petroliferi non possono stabilire però quando il conflitto sarà

compagnie petrolifere delle Nazioni della coalizione. L'Italia, pur essendo la Nazione più vicina al conflitto e pur essendo direttamente coinvolta dall'inarrestabile flusso migratorio, non sembra essere ancora orientata in modo netto e coerente. Va detto, però a chiare lettere che la nostra preoccupazione è rivolta al popolo libico e ai tanti giovani che vedono nell'Italia e nell'Europa un'oasi di democrazia e di libertà, oltre che una risorsa per assistenza e solidarietà. Per quanto riguarda le esitazioni del nostro Paese e il rischio che la nostra politica estera debba essere condizionata dalla netta chiusura della Lega Nord verso gli immigrati, è chiaro che il nostro punto di riferimento deve essere la risoluzione dell'ONU e, di conseguenza, la risoluzione che abbiamo sottoscritto e che è già stata approvata dalle Commissioni parlamentari

altri paesi europei; a monitorare con attenzione e costanza l'evolversi delle previsioni della Risoluzione n. 1970 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU che, ai punti 4, 5, 6, 7, 8 demanda alla Corte Penale Internazionale di aprire un fascicolo di indagine su Gheddafi ed altri appartenenti al Governo libico, per verificare la sussistenza di eventuali crimini contro l'umanità perpetrati nel corso delle operazioni militari,

l'incolumità della nostra popolazione, a cominciare dalle Regioni meridionali, e prevenire, con appositi interventi di *intelligence* le eventuali ritorsioni del dittatore libico. In conclusione, ringrazio i ministri La Russa e Frattini per i loro interventi anche se

del comando, che deve essere affidata, ovviamente, alla NATO; il secondo è la gestione del tema immigrazione, considerato in senso lato.

Va ricordato innanzitutto che la materia immigrazione, nel contesto normativo europeo, circa l'aspetto dell'accoglienza è sì lasciata ad ogni singolo Stato ma, come è stato evidenziato, tra l'altro proprio ieri, in in Commissione affari esteri del Senato, e ricordato dal presidente Dini, l'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea indica proprio il principio di solidarietà, e non solo: indica anche il principio di equa ripartizione della responsabilità anche sul piano finanziario fra gli Stati membri proprio in materia di immigrazione.

Da sempre - ricordiamolo, non fa male, è corretto - il ministro Maroni ha sostenuto questo, ricordando proprio il principio di solidarietà. Oggi ci troviamo evidentemente in un momento di piena emergenza. qualche mio collega ha ricordato alcuni numeri: 15.000 clandestini in tre mesi. La presidente Bonino ha sdrammatizzato

che l'Unione europea deve comunque assumersi. Perché siamo uniti, siamo Europa, ma solo per dividerci gli onori, o siamo uniti e siamo Europa anche per dividerci gli oneri? È questa una domanda alla quale evidentemente chiediamo una risposta ed un impegno da parte del Governo. Il lavoro del Viminale, in un contesto di forte emergenza ed eccezionalità, prosegue. Va però comunque chiarita la distinzione fra profughi e clandestini ricordando che, per quanto riguarda i clandestini, essi troveranno un percorso -ovviamente è previsto - che passerà per i centri di identificazione e di espulsione. Quindi, abbiamo il territorio che, seguendo anche il principio di solidarietà, sta facendo la propria parte, e così dovrà essere anche per l'Unione europea. Il 21 marzo, l'altroieri, vi è stato il primo atto ufficiale da parte dell'Unione. È come è stato ricordato prima dal collega della Lega Nord Divina:

di quegli Stati membri più direttamente interessati dai movimenti migratori, oltre all'impegno a fornire il sostegno necessario.

ricordata all'Unione europea l'importante azione di pattugliamento nelle acque del Mediterraneo in funzione di deterrenza e contrasto alle organizzazioni criminali e terroristiche, ovviamente (e a quelle legate al traffico di esseri umani, altrettanto ovviamente), ma anche in funzione di prevenzione migratoria. Altro impegno proposto all'interno della proposta di risoluzione di maggioranza è quello di ottenere da parte dell'Unione europea un apporto di mezzi, anche finanziari, per condividere l'onere di gestione degli sbarchi di immigrati, essendosi essendosi l'Unione europea, come prima ricordato, impegnata a fornire con prontezza il supporto necessario in base all'evolversi della situazione di crisi.

teso a ridistribuire la presenza degli immigrati tra tutti i Paesi membri, fornendo assistenza adeguata anche alle operazioni di riconoscimento e identificazione di coloro che si dirigono verso le coste italiane. PRESIDENTE. Senatore Alberto

vale l'impegno e fa primeggiare tutto il nostro Paese rispetto a tale questione. Se l'Italia merita la solidarietà da parte dell'Unione europea, ovviamente Lampedusa la deve avere dal nostro Paese; l'avrà ora nell'emergenza grazie all'impegno del Governo, e del Viminale in modo particolare, e alla compartecipazione delle Regioni in proporzione. che questo è il lavoro nell'emergenza. Lampedusa dovrà avere un equo risarcimento per i danni che il turismo e ogni attività locale hanno dovuto subire in questo periodo, oltre che per i disagi che ogni cittadino ha patito. Non sarebbe male quindi spingere tutti insieme una legge *ad hoc*, come più volte evidenziato dalla senatrice Maraventano, facendo in modo che possa essere concretizzata. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli

nel quale gli obiettivi sono chiari: difesa dei civili, senza fare eccezione anche dei mezzi, e aiuto umanitario. Ha lasciato nel barocchismo più pieno gli strumenti perché tra l'altro - e ricordo certamente bene - mette insieme la possibilità dell'intervento dei

non avevano valutato il discorso del ruolo di certezze in una situazione in cui si usa anche la forza, finalizzata in quel modo, come è a tutti noto;

e probabilmente non si fermerà attorno alla questione di Gheddafi; in questa grande realtà che va dall'oceano Atlantico a quello Indiano il problema è per noi importantissimo. C'è un mondo che dà segni di smuoversi da una chiusura che lo teneva in condizioni di centinaia di anni fa. La fragilità di Stati come l'Egitto,

perché chiede più giustizia, il miglioramento delle condizioni di vita, una condizione giovanile più accettabile e il paragone con il mondo oggi è veloce e non lo cancella più nessuno.

NATO. La partita non è chiusa perché la risoluzione dà la possibilità ad uno Stato che voglia comunque intervenire richiamandosi all'utilizzo dei mezzi possibili, anche di spingere la situazione. Bisogna tenere gli occhi aperti, andare avanti, tenere ferma l'attività di coordinamento della NATO. C'è un discorso da aprire sull'Europa:

questa situazione così come si è creata e come si è evoluta, innanzitutto non si è utilizzata la riunione di Parigi per dire che l'Italia voleva svolgere un suo ruolo

l'assistenza logistica, e poi alla fine dire che noi teniamo da parte i nostri mezzi è una furberia che non può essere accettata da chi combatte in ogni modo.

perché, tra l'altro, quello - per chi lo conosce - è un mondo dove queste cose contano più di quanto contano tra di noi. Questa è la raccomandazione che voglio fare che si basa su queste due considerazioni. I nostri interessi passeranno attraverso un'attenzione seria e uno sforzo di comprensione e di aiuto a tutto questo mondo che certamente non

Signor Presidente, colleghi, signori del Governo, a dispetto di tanti profeti di sventura, la maggioranza si appresta a dare oggi in quest'Aula una prova di compattezza. Ringraziamo l'Esecutivo per la sensibilità nei confronti del ruolo del Parlamento, che in altre analoghe occasioni non fu mostrata da quella parte politica che oggi ha ritenuto di polemizzare anche su questo aspetto. Giungiamo a questo appuntamento con una risoluzione unitaria della maggioranza, che impegna il Governo a condurre la sua azione, tenendo ben saldi allo stesso tempo il rispetto degli impegni verso la comunità internazionale e la tutela degli interessi dell'Italia. Nell'auspicare fin da ora che le opposizioni sappiano far prevalere il bene della Nazione sulla facile rendita di una polemica di parte, diciamo con chiarezza, presidente Marini, che ci rifiutiamo di guardare alla crisi libica dal buco della serratura delle dinamiche interne alla politica italiana, come se il frangente che stiamo attraversando consentisse di essere piegato all'esigenza di colpire questo o quell'avversario. Il momento richiede ben altra consapevolezza. Presidente, colleghi, signori del Governo, quando il mondo era diviso in due blocchi, le politiche europee - quelle dei Sei, per intenderci - erano una variabile del quadro internazionale. I margini di autonomia dei singoli Paesi erano ristretti; si agiva soprattutto cercando di influenzare l'Europa in senso più o meno atlantico. In quegli anni, per opera di uomini come Fanfani, Gronchi, Mattei, l'Italia tentò più volte di svolgere una politica autonoma nel Mediterraneo, soprattutto sul versante energetico. Il nome di quella politica Il nome di quella politica fu "neo-atlantica" per il suo collocarsi al confine, e a volte addirittura oltre il confine, tra la legittimità e l'eresia. Da allora il mondo è cambiato. L'Europa si è sempre più allargata, l'asse franco-tedesco è saltato e gli Stati nazionali hanno recuperato una concezione originaria della politica estera, piuttosto che devolverla interamente a un continente che ancora in questi giorni - dico purtroppo - ha mostrato tutte le sue difficoltà a interpretare un indirizzo unitario. In questo nuovo contesto la politica estera del centrodestra ha saputo coniugare il rispetto di un atlantismo non a corrente alternata, incurante del fatto che alla Casa Bianca vi fosse George Bush o Barack Obama, con una strategia di attenzione verso il Mediterraneo. Una strategia che, grazie anche ai buoni rapporti con la Russia, potesse consentire di arrivare laddove in altre epoche altri uomini si erano dovuti fermare, facendo passi in avanti lungo la strada dell'indipendenza energetica e chiudendo pagine tristi della nostra storia nazionale. Perché vedete, cari colleghi, non si può essere politicamente corretti a giorni alterni. Bisognerebbe evitare di essere politicamente corretti, ma quanto meno, se lo si è, Non si può un giorno festeggiare i centocinquant'anni dell'Unità d'Italia e il giorno appresso dimenticare che il nostro Paese fu protagonista di una brutta pagina di pagina di colonialismo già a partire dal 1911, ragion per cui chiudere quel capitolo con atti di riconciliazione per noi era comunque un obbligo, anche di carattere morale. Non si può dimenticare neppure quello spartiacque epocale che è stato l'11 settembre 2001, e il recupero di Gheddafi al fronte anti-terroristico che indusse tutti gli Stati europei, a cominciare proprio dalla Francia e dalla Gran Bretagna, a compiere gesti distensivi nei suoi confronti, e che spinse Romano Prodi, presidente allora della Commissione europea, a dichiarare: «Lo dico con chiarezza: sono stato io a sdoganare Gheddafi, a iniziare l'attenuazione del suo isolamento internazionale. Lo feci quando mi fu chiaro (e le informazioni in mio possesso si rivelarono esatte) che il colonnello stava mettendo da parte la politica di tensioni, guerre e inquietudini che fomentava nell'Africa subsahariana».

pur senza augurarselo, che al mondo diviso in blocchi sarebbe seguito uno scontro di civiltà, e dall'altra evidenziò senza alcun riflesso ideologico, ma come constatazione di fatto, l'incontenibile tendenza all'espansione della democrazia nel mondo. Queste interpretazioni mettono in evidenza la cifra drammatica di questo secolo - di questo primo decennio del secolo - ovvero la coesistenza di due tendenze storiche in conflitto fra loro: da una parte il rischio di sbocchi integralisti, dall'altra la spinta verso processi di democratizzazione e di libertà. Purtroppo non è possibile dividere con una linea netta queste due tendenze, come pure qualcuno vorrebbe. Né si può dividere con una linea netta il bene e il male, valutando delle dinamiche del mondo solo i rischi, o privilegiando solo le opportunità. Gli scenari con i quali ci confrontiamo non sono esenti da chiaroscuri, e per questo chi ritiene che si possa agire oggi al riparo da ogni contraddizione e in nome di un principio di coerenza tanto astratto quanto assoluto si pone fuori dalla storia e insegue certezze fittizie invece di perseguire l'intelligenza - nel senso letterale - e la comprensione di quanto sta accadendo. Ed è esattamente su questa dicotomia che si colloca il dibattito che ha segnato la situazione nordafricana e in particolare la crisi libica. Signor Presidente, colleghi senatori, signori del Governo, la nostra risoluzione si fa carico responsabilmente della drammatica contraddizione dei tempi e degli avvenimenti. Non propone una semplificazione manichea. Corona un percorso di serietà che si addice alla serietà dei tempi che stiamo vivendo. Il testo che la maggioranza offre alla discussione del Senato è il frutto di un approfondimento ulteriore della situazione rispetto alla deliberazione delle Commissioni congiunte. Questo approfondimento ha consentito alla maggioranza di presentarsi oggi convintamente e consapevolmente unita, chiarendo anche quei punti di sospensione che l'urgenza della situazione aveva determinato. Nel merito, non possiamo non rilevare come alcune delle nostre istanze stiano già divenendo tema di attuale realizzazione. Cito ad esempio - l'ha fatto il ministro Frattini la richiesta di attribuzione di un ruolo centrale alla NATO, che l'America sostiene e per la quale la posizione della stessa Francia sta creando condizioni favorevoli. Noi riteniamo che non ci si possa tirare indietro rispetto a un impegno internazionale frutto di un lavoro diplomatico intenso, che ha prodotto la non scontata rinuncia di Russia e Cina all'esercizio del potere di veto e la non contrarietà della Germania, anch'essa non scontata. E, per rispetto della comunità di cui l'Italia fa parte, non possiamo non sottolineare di quale strumento innovativo e moderno l'ONU abbia inteso dotarla, dando corpo, forza e un nuovo orizzonte al principio del mantenimento della pace e della sicurezza nel mondo, lontano dagli stilemi pacifisti che pure per tanto tempo avevano albergato a sinistra. *(Applausi dal per il nostro Paese mostrarsi defilato o addirittura assente nel momento in cui gli equilibri del Mediterraneo vengono messi in discussione Ma se affermiamo che sarebbe suicida, lo facciamo proprio in nome di quegli stessi interessi nazionali che al nostro Paese impongono di adottare un *surplus* di prudenza, di evitare fughe in avanti, di pretendere dai *partner* europei una assunzione di responsabilità. Ce lo chiede la nostra storia. Ce lo chiedono i nostri interessi. Ce lo chiede la nostra posizione geopolitica. Su questa strada ci auguriamo che anche l'opposizione possa convergere. Se non lo farà - lo dico senza alcuna strumentalità - ci auguriamo almeno che spieghi il perché. Che dimostri insomma un interesse effettivo a questo dibattito e non dia neanche l'impressione di voler piegare un tema così importante a esigenze domestiche, a evidenziare divisioni nella maggioranza che non ci sono, perché questo non le farebbe onore.

credo che esse contengano i punti chiave che possono permettere davvero di rinnovare un appello

dalle Commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato, potrebbero essere davvero la sintesi più completa di una posizione nazionale su questa complessa vicenda. Esprimo, con riferimento alla proposta di risoluzione n. 1, parere favorevole del Governo e mi permetto di formulare al senatore Gasparri e agli altri firmatari

la possibilità di «adottare ogni iniziativa per assicurare la protezione delle popolazioni», il riferimento all'informazione costante al Parlamento, che nella proposta di risoluzione n. 1 in verità non c'è,

che dica: «Il nostro Paese che, in un primo momento stava fornendo un importante supporto logistico attraverso la messa a disposizione di ben sette basi militari». Questo «ben sette basi militari» introduce un sindacato di merito su una scelta del Governo che è stata tecnica e fondata su ragioni militari. Ma soprattutto,

Onorevoli senatori, il Governo non può prevedere la sospensione immediata, perché la sospensione è scattata di diritto ed è diventata operativa nel momento in cui la risoluzione n. 1973 è stata adottata; non possiamo «prevedere»: dobbiamo solo prendere atto che il Trattato di diritto è sospeso. O si riformula così, oppure chiedo di comprendere che le mie dichiarazioni hanno chiarito quale sia lo stato giuridico di questo Trattato

che in sostanza non vedrei come negative, ma non possono essere affrontate nel contesto di una risoluzione che riguarda materia del tutto diversa. Esprimo per questo parere contrario sull'ultimo capoverso

nel capoverso che inizia con «se, viceversa, le truppe di Gheddafi persevereranno nell'attaccare sistematicamente le città» si dice: «la comunità internazionale dovrà assumere nuovi e più stringenti impegni per evitare il perpetuarsi di crimini». Chiedo al senatore Rutelli e agli altri presentatori:

onestamente il Governo oggi non è minimamente in condizione di accettare un'ipotesi del genere. Vorremmo chiarire cosa avevano in mente i presentatori parlando di nuovi e più stringenti impegni.

dal Regolamento europeo, che rende inesigibili, da parte degli imprenditori italiani, le prestazioni contrattuali fino a che l'embargo non sarà revocato.

di procedere nel più breve tempo possibile all'adeguamento delle norme interne. Mi permetto di dire, senatrice Bonino, che lei nel suo intervento ha detto qualcosa che il Governo non condivide affatto, affatto, cioè che se il presidente Bashir o il colonnello Gheddafi venissero in Italia non potrebbero essere arrestati. le istituzioni internazionali per pensare di far credere che lo Statuto di Roma non sia già ora immediatamente vincolante per l'Italia, anche senza le norme interne. Questa è giurisprudenza assolutamente pacifica. Noi avremmo l'obbligo assoluto già ora di arrestare persone con un ordine di cattura della Corte penale internazionale. Quindi, non è per questa ragione che reagisco alle sue affermazioni, ma perché è già ora in vigore per l'Italia quest'obbligo. Ciò detto, il Governo si impegna ovviamente ad accelerare, perché è giusto, l'adeguamento delle norme integrative interne.

essendovi già questa sospensione, l'espulsione danneggerebbe il futuro Governo libico, che noi vogliamo arrivi rapidamente nella democrazia. Dunque anche su questo punto, per queste ragioni, esprimo parere contrario. Per il resto, esprimo parere favorevole.

Presidente, in punto di procedura, sarà francamente un mio limite, ma io non ho mai ascoltato

di esprimere il voto sulla proposta di risoluzione n. 2 nella sua interezza, perché è evidente che il testo complessivamente valutato di quella proposta di risoluzione non è la stessa cosa che trasfondere quel testo

dico quali parti accolgo delle modifiche che lui ci propone, restando inteso - se è d'accordo anche la maggioranza - che le parti che intendiamo mantenere verrebbero votate per parti separate. Una parte delle modificazioni vengono quindi accolte,

al più presto possibile l'apertura ai voli civili dell'aeroporto di Trapani

Signor Presidente, mi rivolgo a tutti i Gruppi parlamentari e al ministro Frattini, che è stato con noi oggi durante il dibattito. Credo che dovremmo prendere molto sul serio l'occasione odierna; noi l'abbiamo fatto sin dal primo momento, chiedendo che fossero le Assemblee del Senato e della Camera a valutare

importante e serio, ha riguardato una decisione che nessuno di noi ha assunto con superficialità, ma, al contrario, valutando la pesantezza e la complessità della questione che andava che andava a dirimere e della situazione nella quale andava a inserirsi, quella di oggi ed anche quella di domani. Ma noi rischiamo di concludere questo dibattito con una serie di voti incrociati, per parti separate *(Applausi dal di risoluzione, quella dei colleghi della maggioranza, che mi permetto di definire ambigua e in parte smentita su punti anche cruciali dalle stesse dichiarazioni del ministro Frattini. di chiudere questa discussione con una serie di voti alla fine dei quali anche gli addetti ai lavori avranno difficoltà a rintracciare il filo, la decisione, il senso con il quale il Parlamento si è espresso su una questione così importante per l'Italia, per il suo ruolo, per il suo onore e per la sua credibilità internazionale. Mi permetto, pertanto, sapendo che chiederò a ciascuno di noi, a cominciare da me e dai senatori e dalle senatrici del mio Gruppo, di rinunciare a qualcosa, di concludere questo dibattito votando tutti insieme una risoluzione semplicissima che dica: udita la relazione e le conclusioni del ministro Frattini, le approva.

per confrontarci su una serie di questioni e su un problema che per ammissione di tutti è complesso, soprattutto perché siamo in una fase evolutiva della situazione: domani si terrà un importante Consiglio europeo che tratterà questo tema insieme ad altri,

sia forte nello scenario europeo ed internazionale, essendo il primo Paese coinvolto dalla vicenda libica. Presidente, questo dibattito era iniziato con l'affermazione politica, che accetto come sfida e come constatazione, che la maggioranza non avesse numeri e posizioni. redatto un documento come maggioranza (non avevamo alcun dubbio sulla coesione della maggioranza) e riteniamo corretto porlo in votazione. Peraltro, ribadisco che recepiamo integralmente la proposta di risoluzione

c'è, si assume le sue responsabilità, ma dialoga e si confronta con le vostre proposte, che abbiamo deciso di recepire integralmente.

ho molto rispetto per la proposta avanzata dalla presidente Finocchiaro, che non conoscevo (niente di male, ho detto solo una cosa fattuale). Pensandoci, però, credo di non potervi aderire,

Se la vostra non è una posizione strumentale, non c'è motivo di dire no a questa proposta.

niente e senza una votazione assai complessa, il cui esito non si capisce, conviene sulle dichiarazioni che sono state rese in quest'Aula dal rappresentante del Governo ministro Frattini. Se non è così, la proposta di risoluzione che abbiamo già presentato, e che riproduce il testo che è stato votato all'unanimità, con esclusione della Lega, dalle Commissioni congiunte esteri e difesa benissimo riproduce esattamente lo stesso effetto. Dopo di che, è ovvio che se lo spirito che ci anima non è identico, non possiamo arrivare ad identica conclusione.

auspico più di lei. Avrei sostenuto anch'io l'ipotesi di un voto corale ed unanime del Parlamento sulle dichiarazioni del Governo, ma ogni parte politica è legittimata ad assumere le proprie posizioni, e non sta al Presidente del Senato imporre scelte.

senza né vincitori né vinti, ma con un messaggio unitario al Paese. Questo è il mio interesse di Presidente del Senato, e credo sia l'interesse ed il desiderio di tutti voi. *(Applausi

I Gruppi di maggioranza provvedano come ritengono, dopo aver ascoltato il Governo, a riformulare la propria risoluzione; noi non abbiamo strumenti per impedirlo.

ad esprimere un parere subordinato all'integrazione di una risoluzione con un'altra risoluzione. È un pasticcio! Quindi, la maggioranza si assuma le sue responsabilità. Non si è mai visto - mi permetto di